In queste ore tutti noi che amavamo la sua arte cerchiamo di descriverlo nel modo più fedele e rigoroso possibile. A me colpiva e colpisce quella descrizione minimalista che lui faceva di se stesso in un *blog* che teneva su un noto quotidiano *on line*; si definiva compositore, cantante e regista. Negli anni Settanta, con la sua musica di ricerca, ha attraversato le avanguardie europee e alla fine degli anni Settanta è passato alla musica di larga comunicazione, alternandola a opere classiche. Diceva questo di se stesso. Era un artista davvero poliedrico, che spaziava dalla musica, al cinema (regista di diversi film), alla pittura. Amava muoversi tra i generi musicali più diversi: dalla musica sperimentale e di avanguardia a quella colta, al pop, alla musica elettronica ed etnica, all'opera lirica. Il grande successo e la notorietà arrivarono quasi per scommessa - come raccontava lui stesso - per aver raccolto una specie di sfida lanciatagli da alcuni giornalisti musicali, secondo i quali non sarebbe stato capace di scrivere canzoni popolari. Mai previsione fu più sbagliata, ovviamente, perché Franco Battiato cominciò a scrivere delle canzoni popolarissime, ma mai banali, ognuna delle quali era un gioiello fatto di note che si intrecciavano con parole, pensieri e concetti coltissimi, come mai nessuno prima aveva fatto, segnando una strada compositiva assolutamente nuova. I suoi testi erano assolutamente originali e complessi, impossibili da dimenticare e nei quali mescolava tutta la sua cultura, il gusto per la ricercatezza, il misticismo e l'esoterismo. Arrivarono i successi de «L'era del cinghiale bianco» e, poi, quello fragoroso de «La voce del padrone»: un successo talmente grande che, oltre a lusingarlo per aver vinto pienamente la sfida a cui facevo accenno poc'anzi, in qualche modo lo imbarazzava. Negli anni a seguire continuò la sua ricerca musicale e artistica verso atmosfere diverse e introspettive, donandoci altri capolavori assoluti che hanno segnato la storia della musica italiana e mondiale. Amava coltivare anche collaborazioni con altri artisti, ad alcuni dei quali (specie importanti voci femminili italiane) ha regalato sue canzoni indimenticabili e ha sostenuto e aiutato con la sua generosità Oltre agli ambiti musicali, Battiato - come dicevo poc'anzi - ha percorso altre vie artistiche. È stato regista di diversi film, tra cui uno su un celebre compositore - Beethoven - e anche pittore di opere figurative su tele e tavole,

dei lavori dell'Assemblea ce lo impongono. Voglio concludere affermando che Battiato, in tutta la sua vita, ha coltivato l'arte e la spiritualità, senza abbassarsi a compromessi e rimanendo coerente e rigoroso con se stesso e con i propri principi. Addio maestro, addio compagno delle nostre vite. Eri sofferente da tempo, ma adesso, come cantavi ne «La cura», ti solleverai dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore e guarirai da tutte le malattie.

decidere di essere musicista come Franco Battiato mette di fronte a tante responsabilità, perché è come stipulare un contratto dove vengono elencate tutte le condizioni. Farlo significa avere anche una straordinaria passione, che è la forza motrice per avviare la propria carriera musicale. È un fuoco che arde dentro e non si spegne mai. È voler intraprendere con fermezza un percorso di cui se ne ha consapevolezza già nei primi anni della propria vita. Significa perseverare anche nelle difficoltà, perché si vuole arrivare a un traguardo che ci si è prefissi. E soprattutto vuol dire saper valorizzare il proprio talento, che è fondamentale, anche se non è l'unico fattore determinante. Anche l'essere fortemente motivati nasce dentro in modo naturale e non si affievolisce mai nella vita, come pure la determinazione, che è un'arma potente che si deve saper usare non a discapito degli altri, ma per un uso personale. Essere musicisti, come lo è stato Franco Battiato, significa lavorare sodo ogni giorno; essere produttivi ogni giorno; alternare la teoria della musica alla pratica; prepararsi, dedicarsi appieno alle attività che servono per far sì che la musica diventi tua per sempre, con costanza. E la differenza la fanno i singoli giorni. Pochi minuti, mezz'ora o un'ora al giorno possono sembrare niente, ma nella somma di mesi e anni fanno una grande differenza. Franco Battiato raccoglieva in sé tutte queste necessarie qualità: passione, perseveranza, talento, motivazione, determinazione, preparazione e dedizione. Con innata sobrietà, ma anche con forza ed estrosità ha amato la musica in tutte le sue curve e spigolature, con dolcezza e asprezza, ma sempre con eleganza. È stato il musicista di tante età, abbracciando con le sue creazioni intere generazioni, rigenerando se stesso e la sua musica a tempi ed esigenze diverse. Grazie Franco per aver dato pienezza e senso alla difficile vita dei musicisti; per avere colorato con la tua musica tanti dei nostri giorni; per aver amato e curato fino all'ultimo istante di vita il tuo raro talento. Adesso hai trovato il tuo centro di gravità permanente. Riposa.

grazie a tutti un genio che ha vissuto nella costante ricerca di forme artistiche nuove da sperimentare. «Sono sempre in cammino» spiegava e cantava «l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè. Mi rende schiavo delle mie passioni». Ha avuto sempre un pizzico di autoironia e una tensione creativa costante, che lo ha reso autore di quella musica che è stata colonna sonora dei nostri anni più belli. «La stagione dell'amore viene e va. All'improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni. Perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai». Amava cantare danzando sul palco in un inno alla vita e all'amore, motore di tutte le cose. La passione carnale è raccontata in «Sentimiento nuevo» e il desiderio di spiritualità per comprendere appieno l'essenza dell'essere umano cantato nella celebre «E ti vengo a cercare». Racconti lirici, riferimenti filosofici e letterari dal sapore antico inseriti in brani dal gusto pop hanno conquistato intere generazioni grate a questo artista unico. il mondo classico e le filosofie orientali, la curiosità verso culture lontane, l'esotismo e poi la Sicilia - la sua e la mia Sicilia l'amore e il dolore per una terra complicata e intensa, ricca di storia e cultura, coraggio e contraddizioni, il mare e il fuoco in un'esplosione di emozioni. L'attrazione verso il mondo della natura si percepisce nella celebre «Gli uccelli», che ha la potenza di farci sentire la libertà e l'emozione di voli imprevedibili imprevedibili ed ascese velocissime «nello spazio, tra le nuvole, con le regole assegnate, a questa parte di universo». E poi la speranza in una società più attenta alle ragioni dell'altro: «Sogno il dialogo con chi la pensa diversamente da me», confidava. Non mi soffermerò sulla breve parentesi del suo impegno politico: oggi voglio ricordare il cantautore, il compositore, il direttore d'orchestra che ha scandito i miei anni magici e irripetibili; anni che probabilmente non sarebbero stati così speciali senza la sua musica. Per sempre grazie di tutto questo, maestro.

chissà se a Franco Battiato avrebbe fatto piacere la commemorazione in suo onore e memoria che stiamo svolgendo qui, in quest'Aula parlamentare, schivo e riservato com'era. Lui che pare non gradisse neanche essere chiamato maestro. La sua parola più eloquente il silenzio: «Dovremmo metterci tutti in cammino come lui, per trovare la bellezza», sono state le parole del sacerdote che ha celebrato ieri i suoi funerali. In un mondo di eccessi, soprattutto di eccessi di parole, di chiacchiere a profusione, Battiato ha insegnato che ciò che conta è l'essenziale. Lo ha fatto nel corso di decenni di attività artistica, passando dalla ricerca musicale sperimentale fino al *progressive* rock*,* dal pop commerciale alla lirica, con la particolare alchimia dei suoi testi, tra suggestioni linguistiche, echi dell'anima, viaggi a volte quasi onirici che ci hanno trasportato nei suoi mondi immaginifici. E poi Franco Battiato ha portato nella canzone il misticismo, la spiritualità, l'idea di un alto, di una linea verticale che, opponendosi alla sola orizzontalità della vita terrena, ci spinge verso lo spirito. In un momento per l'intera umanità come questo, intriso di dubbi e incertezze sul futuro, e con un presente che cerca di scrollarsi di dosso il peso di un evento assurdo e imprevedibile nella sua gravità come la pandemia che stiamo attraversando, il messaggio che ci lascia in eredità Franco Battiato ci arriva forte come un testamento e lieve come una carezza; forte nella spiritualità che Franco Battiato ha coltivato fino alla fine, con la sua fede solida e viva come l'Etna della sua terra, la Sicilia, dove scelse di vivere e di morire; e lieve, come la carezza de «La cura», uno dei suoi brani più significativi, espressione della sua umanità generosa e responsabile del bene verso gli altri. Ed è proprio questo, in questo momento, il testimone da cogliere per le nostre vite, nel nostro operare, nel rapporto con gli altri, con chi incontriamo nelle nostre giornate. Ricordiamoci di togliere la maschera, non quella della protezione dal virus, ma quella che crediamo debba proteggerci dal nemico che temiamo esserci nell'altro, e abbiamone invece cura, per quanto possiamo. Grazie, Franco Battiato!

credo che Franco Battiato avrebbe sorriso molto delle nostre parole, di questa commemorazione in Aula perché la traccia dell'ironia è stata la chiave di tutto il suo percorso artistico. Lo è stata perché i grandi intellettuali, i grandi artisti, i grandi uomini di cultura riescono a compiere un cerchio e padroneggiano talmente tanto l'enormità delle letture e delle riflessioni che hanno affrontato nella vita che, a un certo punto, sono in grado di trasformarle in quella parola, in quella musica, in quella nota che possono sembrare di una semplicità inaudita, che possono sembrare uno scherzo, un gioco per qualcuno, quando in realtà sono esattamente quel ponte che permette a chiunque

la straordinaria dimensione popolare stia proprio qui, in una continua sfida innanzitutto con sé stesso, ma anche con il suo lettore, con il suo ascoltatore, dal punto di vista sia musicale

per provare a vedere se dentro a quella parola, a quella citazione, a quella evocazione c'era qualcuno che stava al gioco e provava ad andare a vedere che cosa si voleva raccontare davvero. Così, nelle parole di Battiato, si attraversavano le epoche e i territori. Ha portato l'Estremo Oriente; oggi questo è molto più consueto, ma l'ho fatto molto prima; ha portato la nostra fondamentale relazione con l'altra sponda del Mediterraneo e con il mondo arabo. Del resto chi, se non uno straordinario siciliano, avrebbe potuto fare questo. Ci ha portato le culture e le religioni diverse: l'induismo, il buddismo, i mistici, la filosofia, la grande filosofia greca; ci ha fatto cantare versi di Eraclito andando ad approfondirli e a coglierli con una profondità che gran parte delle letture filosofiche scolastiche magari non affronta nemmeno, perché, certo, tutto scorre, ma soprattutto a passare invano è il vero senso della vita. Questa è la grande lezione di Eraclito ed è anche la grande lezione di passaggio in quell'album meraviglioso che è «L'imboscata». Poi ha detto molto alla politica. Lo ha fatto in prima persona come cittadino impegnato, ma anche attraverso le sue canzoni e ha sempre tenuto insieme questi due elementi, perché tutti ricordano gli anni de de «La voce del padrone», la scelta di diventare pop e di quegli anni ricordano «Bandiera bianca», ricordano quel suo razzismo che lo teneva lontano da programmi demenziali con tribune elettorali. sono cresciuti molto nella nostra società e le tribune elettorali oggi noi le rimpiangiamo, perché erano dei luoghi di approfondimento rispetto a quella che è la politica in televisione oggi. Questo Battiato ce lo ha ricordato tante volte, ma non per tenersi lontano dall'impegno politico, ma per avvicinarsi con profondità, per non essere quelli che cambiano le maglie ogni volta che cambia la stagione; per non essere quelli che si innamorano del potere; per essere quelli che invece si appassionano della sofferenza degli uomini e delle donne in ogni parte del mondo, che si ricordano dei migranti che cercano una speranza per la propria vita, come nell'ultimo meraviglioso pezzo che incrociava insieme il senso

si sia trasformato: lui, infatti, credeva nella reincarnazione, temeva di potersi incrociare in una formica o in un serpente. Credo che non sia così così e tornerà in tante forme e sarà presente in mezzo a noi con le sue parole, con le sue note, con le sue musiche e noi dovremmo saperlo ricordare con le nostre azioni in quest'Aula. oggi ricordiamo la figura di Franco Battiato, catanese, cantautore eclettico, artista dal linguaggio emotivo capace di evocare, senza mediazioni, le voci del cuore. È questo ciò che rimpiangiamo oggi: non il personaggio che si avvicinò alla politica, bensì l'artista, il genio musicale, il filosofo sempre all'avanguardia, alla ricerca di una stabilità che influenzasse l'essere umano, senza far cambiare idea sulle cose e sulla gente, un centro di gravità di cui tutti in questo periodo abbiamo sentito un'enorme necessità. Aveva scelto di stabilirsi a Milo, paese etneo, mantenendo una riservatezza e una semplicità assoluta, partecipando e organizzando numerose manifestazioni musicali durante le estati milesi. Le sue opere rimarranno con noi negli anni a venire e l'omaggio che gli vogliamo rendere è l'impegno a non dimenticare la cura che ci ha donato, attraverso la sua musica, definendoci esseri speciali. Mi preme evidenziare Mi preme evidenziare come alla Camera il collega Mollicone abbia avanzato la proposta di dedicare un istituto culturale a Franco Battiato e come già anche a Catania il sindaco Pogliese abbia proposto e poi deciso di intitolare il lungomare della città al nostro artista catanese. Era necessario intestargli un luogo che ne ricordasse la grandezza artistica, così riferisce il sindaco. Nella mia introduzione ho detto come fosse un artista eclettico per

sembrare un po' dicotomico rispetto al suo orientamento politico, in realtà non è assolutamente Battiato nacque a Riposto, in provincia di Catania - come sapete, quello è anche il mio territorio - ed era visto con molto rispetto. Studiò filosofia all'Università di Catania ed effettivamente il contenuto dei suoi testi testi esprime in pieno la sua formazione e l'attenzione culturale anche al territorio siciliano, che è stato un crocevia di di culture. Non a caso, alcuni testi e video che riprendono le sue creazioni riportano dei collegamenti con la realtà culturale araba. Fratelli d'Italia - come ho esposto - ha già avanzato delle proposte concrete e speriamo che la proposta avanzata anche dalla Camera possa trovare rapido compimento.

Qua e là, ci sono canzoni a cui qualcuno ha avuto la generosità di riconoscere un valore letterario. Erano riconoscimenti liberi dall'invidia e dal livore. Telefonate che facevano piacere». Ma non di solo valore letterario si tratta per le sue canzoni, bensì anche di ricerca esistenziale e direi filosofica e del lascito profondo che hanno donato ad intere generazioni. Sperimentazioni musicali e testi importanti rappresentano il contrassegno della sua opera, come la frase emblematica del «Centro di gravità permanente»: «Gesuiti euclidei Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori Della dinastia dei Ming», che si riferiva al gesuita Matteo Ricci. Le sue opere, infatti, sono intrise dell'incontro tra culture diverse, di contaminazione tra Oriente e Occidente. Occidente. Dalla sua terra alle pendici dell'Etna, una terra vulcanica, ha tratto l'energia necessaria per aprirsi al mondo e alle differenze, ma ha radici ben salde nella sua Sicilia, al punto da portarlo anche a una sperimentazione politica, proprio lui che aveva speso parole durissime all'indirizzo della classe politica. Proprio dalla comunanza tra terre vulcaniche angoscianti, energetiche e vitali nello stesso tempo, qualche anno fa a piazza Plebiscito il popolo napoletano, generalmente geloso delle sue canzoni, ha applaudito commosso alle note di «Era di maggio» cantate da Franco Battiato. Uomo del Sud, dunque, se n'è andato proprio nel mese di maggio e come recita la bellissima canzone del poeta Salvatore Di Giacomo che Battiato aveva interpretato in maniera dolcissima, fuori dai canoni classici: «Si stu sciore torna a maggio Pure a maggio io stonco ccá» (Se questo fiore torna a maggio anche a maggio io sto qua). Del resto, nella sua ultima opera «Torneremo ancora», dal silenzio delle sue apparizioni pubbliche, egli stesso ha gridato: «La vita non finisce!».

«squisitamente enigmatico non per vizio di vanità, ma per instancabile curiosità, studio e sperimentazione». Così è stato scritto di Franco Battiato e così è stata la sua vita di uomo e di artista. Consentitemi una citazione dai suoi testi sferzanti e poetici: «E ti vengo a cercare Con la scusa di doverti parlare Perché mi piace ciò che pensi e che dici Perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine Saturo di parassiti senza dignità Mi spinge solo ad essere migliore Con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni». Forse riflettere su queste parole è per ciascuno di noi il migliore atto di omaggio che, come parlamentari della Repubblica, possiamo dedicare a Franco Battiato, al suo essere speciale. Grazie Franco Battiato! Abbiamo esaurito gli interventi in ricordo di Franco Battiato. Mi unisco all'elogio della sua musica, dei suoi testi. l'unico che è riuscito a citare un filosofo come Guénon in una canzone Sull'uomo, avete detto voi. **Discussione

noi siamo qui oggi per un passaggio importante per l'agricoltura e per molti territori del nostro Paese. Credo sia una cosa bella il fatto che siamo qui ad approvare al Senato la legge sull'agricoltura biologica a pochi giorni dalla Giornata mondiale sulla biodiversità.

negli ultimi due anni; con una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica; con il cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica; con una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione 3 miliardi di valore del comparto, la crescita continua della produzione dell'Italia e dell'*export* e paradossalmente - finalmente - grazie alla crescita del mercato interno, una riduzione dell'*import* di biologico che avevamo fino a qualche anno fa. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, con il *green deal* europeo e come *farm to fork*, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica. L'Unione europea conta di investire a partire dall'anno prossimo oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa. Tra l'altro, prevede anche, a partire dal 2022, un nuovo regolamento che introdurrà semplificazioni procedurali, un'ulteriore rivisitazione dei controlli, un rafforzamento forte dei controlli del biologico che arriva da Paesi terzi e una semplificazione delle procedure per la certificazione dell'agricoltura biologica. all'interno di un quadro più generale di politiche agricole e ambientali europee che punta alla riduzione del 50 per cento dell'utilizzo di fitofarmaci,

per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro prospettiva, perché senza questo metodo di agricoltura biologica molti territori, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana, non avrebbero nei fatti una prospettiva economicamente sostenibile. Venendo al testo che oggi discuteremo, l'articolo 1 tratta dell'oggetto e della finalità della norma,

All'articolo 5 si prevede l'istituzione di un tavolo tecnico che sovrintenderà all'agricoltura biologica. All'articolo 6 si prevede l'istituzione di un marchio dell'agricoltura biologica nel nostro Paese. All'articolo 7

al metodo biologico e sostenere la costituzione di forme associative che aiutino le imprese agricole; incentivare il consumo di prodotti biologici; monitorare l'andamento del settore, correlando l'effettiva produzione alle superfici che vengono utilizzate per realizzarla; sostenere e promuovere i distretti del biologico; favorire l'insediamento di nuove aziende, soprattutto in quelle aree marginali e montane a cui facevo riferimento prima; migliorare il sistema di certificazione e di controllo; incentivare e sostenere la ricerca promuovendo progetti di tracciabilità, in modo da dare garanzie ai consumatori. All'articolo 8 è previsto un Piano nazionale delle sementi biologiche, sapendo che il tema delle sementi è cruciale per questo tipo di agricoltura. All'articolo 9

All'articolo 10 vi è la previsione di strumenti di integrazione per aiutare la filiera biologica nel suo complesso.

la conversione all'agricoltura biologica e per stimolare un approccio territoriale. È fondamentale per l'agricoltura biologica che non sia un tema di singole aziende, ma un tema di territori. di semplificare l'applicazione delle norme della certificazione proprio a livello di territorio; favorire lo sviluppo e la valorizzazione e la promozione dei processi

Il Ministero e le Regioni sono impegnate in tal senso a rafforzare e promuovere questo sistema di agricoltura. L'articolo 14 disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, tenendo conto dello specifico dell'agricoltura biologica in termini di dimensione e struttura delle organizzazioni professionali. All'articolo 15, parliamo di accordi quadro proprio per rafforzare il tema della filiera. L'articolo 16, disciplina le intese di filiera per l'agricoltura biologica. il tema delle organizzazioni dei produttori agricoli. Viene affrontato tutto il tema del riconoscimento e della disciplina di queste organizzazioni, ridefinendone e caratterizzandole proprio su questo tipo di aziende. All'articolo 18 viene normato tutto il tema della certificazione delle sementi, che ripeto essere un tema fondamentale, proprio perché dentro il mondo dell'agricoltura biologica vi è il tema dello scambio e della valorizzazione di piccole nicchie di sementi particolari, legate al contesto in cui vengono prodotte, che qui viene normato. la delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle normative sui controlli per la produzione agricola biologica, richiesto a gran voce proprio alla luce dell'esperienza maturata in questi anni il decreto legislativo attualmente in vigore. Abbiamo nelle nostre mani una vera e propria legge quadro e noi crediamo che possa mettere in condizione

Paese. Su questa realizzazione ci giocheremo una fetta importante, proprio per il rilevante ruolo di crescita nell'agricoltura che questo settore sta rivestendo. Voglio chiudere con alcune considerazioni per chiarire talune questioni e certi aspetti di cui si è parlato in questi giorni,

e arretrato. L'agricoltura biologica oggi si gioca, invece, su una frontiera diversa, quella dell'innovazione, per ridurre i fitofarmaci,

legate all'agricoltura di precisione, legate ai metodi di intervento meccanici e fisici, al recupero di un benessere complessivo dell'ambiente, delle colture e degli animali. Parlo dell'agricoltura simbiotica, dell'utilizzo del *biochar*, dei distillati di legno e di tanti altri prodotti che si stanno sperimentando. Un'ultima considerazione è legata alla questione del biodinamico. Noi in questa legge ci siamo attenuti ai fatti e i fatti dicono

rappresentante del Governo, colleghi senatori, oggi è la Giornata mondiale delle api, che si celebra il 20 maggio di ogni anno, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano le api e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. ricordare in questa sede insieme a voi, cari colleghi, tutti i nostri apicoltori italiani, che sono oltre 60.000. Si contano un milione e mezzo di alveari, che producono 23 varietà di miele, per un valore per il nostro Paese che supera i due miliardi di euro.

di un atto vandalico che gli ha distrutto 70 arnie e ucciso milioni di api. Mattia, non mollare, noi siamo tutti con te. Vivano tutti gli apicoltori italiani!

Questo disegno di legge, già approvato alla Camera dei deputati, risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre. I dati hanno rilevato una crescita dei terreni agricoli coltivati con il metodo dell'agricoltura biologica e delle vendite al dettaglio dei prodotti biologici. Noi cerchiamo non solo di inquadrare bene dove si inserisce il provvedimento e cosa andrà a regolamentare, ma soprattutto di proteggere e tutelare le produzioni italiane, che sono sempre sotto attacco (ve lo ricordo, cari colleghi). Nel mondo, come è stato detto in precedenza, 72 milioni di ettari sono coltivati con sistemi biologici, comprese le aree in conversione. L'Europa coltiva il 23 per cento di questi territori, circa 16 milioni di ettari. I primi tre mercati globali per vendite sono gli Stati Uniti, con 44 miliardi di euro, l'Unione europea, con 41 miliardi, e la Cina, con 8 miliardi.

in Danimarca, in Svizzera e in Austria. L'Italia è al vertice; è infatti il primo Paese dell'Unione europea, con 80.000 aziende e oltre 2 milioni di ettari coltivati. Come ettari coltivati siamo dietro solo alla Spagna e alla Francia. È anche il terzo Paese dell'Unione europea per mercato interno, con 3,6 miliardi di euro. Un ulteriore fattore in grado di accrescere il settore è rappresentato dalle politiche europee, che si stanno avviando proprio in questi mesi e negli anni a venire: il *green deal*,il *farm to fork*. L'Europa, infatti, si è posta come obiettivo quello di aumentare il numero di terreni agricoli condotti in regime biologico del 25

ed è in grado di attivare imprenditoria giovanile (oltre il 20 per cento dei giovani si sta avvicinando a questo settore) e generare nuova occupazione. È stato varato anche il Piano d'azione europeo per il biologico 2021-2027, che supporta con iniziative concrete gli obiettivi del *green deal* europeo, delle strategie della biodiversità. Si prevedono, infatti, investimenti importanti per il 2021, per oltre 49 milioni di euro, e l'istituzione di appalti *green*, che prevedono l'integrazione dei prodotti biologici nei criteri minimi obbligatori per gli appalti sostenibili, ad esempio nelle mense scolastiche e negli ospedali. Tra le novità normative presenti nel disegno di legge sull'agricoltura biologica vi è l'introduzione di un marchio "bio" italiano, così da distinguere tutti i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate nel nostro Paese: un modo per garantire la massima trasparenza sull'origine e sulla filiera dei prodotti e per rendere maggiormente consapevoli i consumatori. Viene istituito inoltre un tavolo tecnico presso il Ministero delle politiche agricole, che coinvolgerà gli esperti del settore. Viene rafforzata la filiera biologica, attraverso la promozione dell'aggregazione tra produttori. Per migliorare il testo abbiamo inserito un nuovo articolo in Senato, l'articolo 19: in particolare, attraverso lo strumento della delega legislativa, il Governo dovrà provvedere, con l'introduzione di un sistema più trasparente, a risolvere il conflitto di interesse che c'è tra controllori e controllati, a beneficio del mercato e della concorrenza; rafforzare le tutele nei confronti dei consumatori; riordinare la disciplina delle lotte contro le frodi alimentari. Onorevoli colleghi, è stato fatto un ottimo lavoro; probabilmente non è il migliore in assoluto, tutti abbiamo contribuito con il nostro lavoro di confronto con le organizzazioni di categoria, con il settore, con i produttori, con i trasformatori, con i consumatori (che sono importantissimi), a renderlo più efficiente ed efficace possibile. Basta chiacchiere, ci vogliono i fatti. L'agricoltura biologica italiana è tra le eccellenze europee e mondiali. Difendiamo le nostre produzioni con un concetto fondamentale che ci deve guidare sempre, in ogni istante: il consumatore finale è il vero datore di lavoro di tutta la filiera agroalimentare. *(Applausi)*. Signor Presidente, oggi stiamo discutendo un provvedimento che affronto un tema atteso e di grande rilevanza: si parla di disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. legato all'agroalimentare e all'agricoltura soprattutto nella mia Regione, la Sicilia, che punta soprattutto ad un'agricoltura biologica, è sicuramente urgente e necessario. necessario. Molti sono i prodotti che presentano caratteristiche organolettiche che risultano un toccasana per la salute umana: ad esempio, l'olio d'oliva, ma anche il succo d'arancia (da noi, soprattutto il tarocco), il pomodoro, ricchissimi di antiossidanti in grado di allontanare i radicali liberi presenti nel nostro organismo.

Con il biologico si riesce a produrre senza prodotti chimici. La lotta biologica e l'uso di prodotti organici si traduce con metodo bio, che si sposa perfettamente con il concetto di salute legato al prodotto. La produzione biologica ha però dei costi sicuramente maggiori rispetto all'agricoltura tradizionale e deve essere sostenuta da misure in grado di integrare il reddito degli agricoltori. Il nostro territorio è senza dubbio una fabbrica naturale di salute da Nord a Sud. Il biologico è l'unica alternativa per un'alimentazione sana, soprattutto per quanto riguarda la lotta ai pesticidi come il glifosato. A tale riguardo, la Sicilia attesta il suo primato in Italia, secondo il rapporto SINAB. I dati ci fanno ben sperare anche sull'acquacoltura, ponendosi come nuovo baluardo. L'Italia è uno dei principali attori nel comparto biologico grazie all'enorme biodiversità del nostro territorio. Tuttavia, è un valore da custodire e da proteggere con estrema cura e attenzione, a causa della sua fragilità. Per questo motivo bisogna sempre adoperarsi premiando le aziende che garantiscono prodotti freschi e salubri, rispettando il giusto costo del lavoro, lo sforzo e l'impegno di ogni giorno a protezione dell'ambiente, della salute alimentare e della trasparenza.

con una dotazione parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale dovuto dalle imprese titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Tra questi prodotti sono inclusi quelli di cui il codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Innovativa risulta altresì l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Le risorse finanziarie del fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti dal finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e del Piano nazionale delle sementi biologiche, per l'istituzione del marchio italiano, per il finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, per i percorsi formativi e per l'aggiornamento di docenti, previsto già all'articolo 11, in cui si prevede, di operare con un sostegno alla ricerca tecnologica applicata nel settore. altresì interessante l'articolo 12, volto proprio alla formazione professionale del settore, dettando nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di distretto biologico, di organizzazioni interprofessionali, di accordi quadro, di intese di filiera e organizzazioni di produttori biologici. L'articolo 18 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Ritengo si debba ribadire che il numero di regole approvate in sede europea per il settore non risulta in linea anche con i livelli e gli *standard* di qualità applicati in Italia. alle conclusioni, ribadisco l'importanza della manutenzione dei territori, come valida salvaguardia per la prevenzione dei dissesti idrogeologici e per la prevenzione degli incendi, che solo il mantenimento di un'agricoltura ecosostenibile può garantire. Se ci si ferma solo alla produttività in agricoltura, certamente non si tratta di un'attività redditizia, ma se solo allarghiamo lo *zoom* e ne valutiamo gli effetti nell'ampio raggio e nel corso del tempo, l'agricoltura biologica è un saggio investimento. Dobbiamo imparare a considerare le cose in modo sistemico e, come mi piace ripetere da qualche tempo, olistico, giacché tutto è economia.

Daniela Ducato, l'imprenditrice sarda di Guspini che utilizza gli scarti organici per realizzare materiali edili ad alta prestazione tecnologica, una bioimprenditrice, cavaliere della Repubblica e campionessa mondiale di innovazione. Il suo filo conduttore è la lana delle pecore sarde, trasformata in risorsa speciale per l'edilizia e l'agricoltura sostenibili. È sua l'invenzione di un prodotto, costituito da lana di pecora, olio d'oliva e ingredienti di scarto di lavorazioni vinicole, residui di pulizia delle arnie, propoli e miele, riutilizzati a vantaggio dell'ambiente, in sostituzione di diserbanti chimici, che alterano il pH del terreno. Nessun additivo chimico, glifosato o veleni sono contenuti nei diserbanti della Ducato. La funzione erbicida è svolta sfruttando il vapore e il calore. Così proteggiamo gli orti, i vigneti, i frutteti e anche il verde urbano. Così garantiamo la sicurezza ai consumatori e agli agricoltori, assicurando il rispetto del suolo e non ne alteriamo il pH, così introduciamo il biologico. Pensiamo ai piccoli appezzamenti di terreno che si ereditano da padre in figlio, coltivati a vigneto e oliveto, e lavorati da mani sapienti, da chi con passione e sacrificio semina, pota, raccoglie e protegge dagli incendi, diventando custode di quel territorio. La produzione biologica è diventata un'attività con funzione sociale e ambientale, i cui prodotti devono essere accessibili a tutti, perché tutelano la nostra salute e quella degli animali, preservandone l'ambiente. disegno di legge in esame individuerà le strategie per favorire le aziende agricole, che si potranno facilmente convertire al metodo biologico, delineando indirizzi e priorità migliorerà il sistema di controllo e di certificazione per garantire la qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa. Come previsto dalla normativa europea, la certificazione biologica garantisce tutti i livelli della filiera produttiva. Il consumatore si sentirà tutelato, se chi produce e chi vende sarà sottoposto a controllo, con ispezioni serie *in loco*. È da notare come, per la prima volta, una regolamentazione europea consideri la produzione biologica, accostandola alla promozione della qualità alimentare. Punto sostanziale: deve essere osservato ciò che entra nel cibo, dalla coltivazione alla produzione e alla trasformazione, fino ai mangimi destinati agli animali d'allevamento che producono la carne e il latte. Il cibo biologico di qualità per noi sarà sempre quello italiano, di nostra produzione, perché amiamo la cultura e il rispetto delle nostre tradizioni. Noi consumatori italiani vogliamo probabilmente nutrirci soltanto con cibo italiano di qualità, che arrivi sulle nostre tavole dalle nostre coltivazioni e dai nostri allevamenti. Non ci interessano gli alimenti sintetici, modificati, stravaganti; mi riferisco all'Unione europea, che considera le tarme della farina un nuovo alimento da consumarsi essiccato. Anche se non dovesse rappresentare un rischio per la salute e si lasciasse libera scelta al consumatore, credo che il consumo dei cibi legati alla qualità, alla tradizione e al nostro territorio ci garantirà prima di tutto la salute e la longevità. legge prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero delle politiche agricole, che coinvolgerà esperti, ricercatori e rappresentanti della produzione bio, per individuare le criticità e offrire delle nuove soluzioni. L'obiettivo della legge sarà anche quello di rafforzare la filiera del biologico incentivando le organizzazioni interprofessionali e le aggregazioni fra i produttori; ma soprattutto si chiede al Governo di rivedere e riordinare le norme sui controlli e sulle frodi alimentari. Infatti sono le frodi e i pochi controlli che mettono a rischio un mercato in grande crescita. L'Italia è il primo Paese europeo per numero di aziende agricole impegnate nel biologico; quindi ricognizioni di norme e revisione della disciplina sanzionatoria sono indispensabili, qualora si utilizzasse impropriamente il marchio biologico italiano che caratterizza i prodotti bio italiani. Si dia quindi sostegno alla ricerca in agricoltura biologica, per garantire la qualità dei prodotti e la tutela dell'ambiente a salvaguardia della biodiversità.

Signor Presidente, gentili colleghi, membri del Governo, come primo commento generale mi viene da dire che forse ci si poteva o doveva aspettare una legge sull'agricoltura tutta, tutta, che coinvolge 500.000 aziende, e non su un'agricoltura di nicchia, i cui numeri andrebbero veramente spiegati in modo proprio, perché sostenere che il 16 per cento del terreno italiano è dedicato all'agricoltura biologica non spiega quanta di quella percentuale è dedicata a prati e pascoli, che ricevono sussidi, ma non producono alcunché. Quindi bisogna veramente spiegare. Torniamo alla legge. Noto con piacere - lo voglio riconoscere al relatore e alla Commissione - alcune migliorie al testo, che hanno almeno in parte recepito indicazioni e rilievi provenienti dal mondo produttivo e dagli studiosi in ambito agricolo. Sottolineo due migliorie: l'introduzione del nodo dei controlli all'articolo 19 e l'eliminazione del riferimento all'interesse nazionale dall'articolo 1. Rispetto a questo aspetto, ho espresso in più occasioni come non vi sia alcun interesse nazionale in un protocollo produttivo di nicchia i cui prodotti non offrono alcuna garanzia di maggiore salubrità e alcun maggiore apporto nutrizionale significativo, come è scientificamente accertato e come è anche indicato nelle linee guida alla ristorazione del nostro Ministero della salute. In sintesi, si tratta di prodotti che si trovano nei supermercati a prezzi doppi o tripli rispetto a quelli privi di certificazione biologica, ma che non hanno nulla di più se non il prezzo. Ecco perché mi spaventa, seguendo le parole del relatore, che si voglia incentivare il consumo del biologico. Perché? anche viene ristabilito un principio di realtà, rimuovendo il riferimento all'interesse nazionale, ho comunque molti motivi di dissenso su questo disegno di legge. Oggi ne tratto uno, che reputo essere un'abnormità normativa e che in primo luogo, se non affrontato da noi oggi con una meditata riduzione del danno, esporrà quest'Assemblea al ridicolo scientifico. Ho presentato tre emendamenti volti a eliminare almeno il richiamo esplicito e il riconoscimento in via preferenziale a pratiche non solo antiscientifiche, ma schiettamente esoteriche e stregonesche. Mi riferisco all'equiparazione, ai fini del presente provvedimento, tra l'agricoltura biologica e quella biodinamica, una pratica agricola i cui disciplinari internazionali comprendono l'uso di preparati a base - cito testualmente - di letame infilato nel cavo di un corno di una vacca che abbia partorito almeno una volta. Il corno, una volta riempito, viene sotterrato per fermentare durante l'inverno e recuperato nei giorni prossimi alla Pasqua per essere sottoposto alla - cito fondamentale operazione di miscelazione e dinamizzazione con acqua tiepida di sorgente, pozzo o piovana, che ha una durata di circa un'ora e può essere effettuata manualmente, ma anche tramite macchine speciali. Vi ricordo che i bovini non perdono le corna come i cervi; le corna vanno segate dai crani, ma il disegno di legge n. 988 (né - mi sembra - alcun disciplinare) non ci spiega se si deve prima macellare l'animale e tagliare le corna, oppure se queste vanno potate dall'animale ancora vivo. *(Applausi)*. Sarebbe meglio disciplinare questa pratica per evitare abusi. Questo che vi ho appena segnalato si chiama preparato 500 dell'agricoltura biodinamica (detto anche cornoletame). Ascoltate come funziona. Secondo il disciplinare, le corna di vacca catturano, quando la vacca è in vita, i raggi cosmici affinché, quando sarà morta o a corna espiantate, il letame in quei corni, seppelliti e diseppelliti in funzione di combinazioni astrali, riceverà le forze eteriche astrali catturate dalla punta del corno, aumentando così il potere di quel letame quando è disseminato sul campo. Mi sono sempre chiesta quale sarà la dose di raggi cosmici che le corna devono catturare (le vacche devono essere primipare) affinché tutto ciò risulti efficace. Nei preparati dell'agricoltura biodinamica c'è anche il preparato 502, ossia una vescica di cervo maschio riempita di fiori di achillea, lasciata essiccare al sole per tutta l'estate, sotterrata a 30 centimetri di profondità (non un centimetro in più) in autunno e dissotterrata sempre nel periodo di Pasqua. Nello stesso disciplinare del marchio registrato Demeter, una multinazionale con sede all'estero alla quale si pagano *royalty*, si specifica che ogni preparato biodinamico sviluppa una forza potente e sottile, il cui effetto può essere comparato con quello dei rimedi omeopatici, ossia è assolutamente nullo e indimostrabile dal punto di vista scientifico. delle domande. Per le vesciche, di quanti cervi maschi ci sarà bisogno? Una vescica per ogni azienda biodinamica? Esiste una deroga alla pratica venatoria che consenta l'abbattimento di tanti splendidi animali dai nostri parchi nazionali, oppure si pensa di importare dall'estero vesciche urinarie estirpate in altre Nazioni o continenti? Colleghi, rimuovere la parola biodinamica dal disegno di legge, come chiedono i miei emendamenti, non impedisce ai produttori di perseguire queste pratiche e ottenere la certificazione di prodotto biologico (per averla basta rispettare i protocolli), ma esplicitare il riferimento al biodinamico in questo testo di legge avrà l'effetto di dare dignità al cornoletame. Aggiungo anche che si tratta di equiparazioni tra biologico e biodinamico solo per la parte nella quale il biodinamico mima le pratiche biologiche, ma di una totale equivalenza, al punto che il disegno di legge in discussione prevede che una quota di fondi pubblici venga dedicata specificamente alla ricerca scientifica, alla formazione nel settore biologico e, quindi, all'equiparato biodinamico. Se quest'equiparazione

Grazie ai fondi previsti dalla legge si potrebbero creare attività e istituire insegnamenti, con tanto di crediti formativi, sulla profondità migliore a cui sotterrare a cui sotterrare le vesciche di cervo, sulla direzione giusta con cui mescolare il letame o su come meglio orientare la vacca al pascolo perché catturi raggi cosmici. Credo che l'errore nel sostenere tutto ciò derivi da una cattiva lettura di un regolamento UE del 2018, relativo alla produzione biologica, dove compare la parola «biodinamica», ma non per un'equiparazione. È una mera citazione. mera citazione. Due citazioni danno la definizione di preparati biodinamici come miscele tradizionalmente utilizzate nell'agricoltura biodinamica. La terza citazione si limita a dire che è consentito l'uso dei preparati Questa citazione è sufficiente a sdoganare l'esoteria biodinamica nelle leggi italiane. Naturalmente il fine ultimo è creare mercato per prodotti che non hanno alcuna caratteristica superiore superiore scientificamente accertata rispetto a quelli da agricoltura integrata, se non i costi. Continuerò, pertanto, a fare la mia doverosa parte per segnalare in ogni occasione che i prodotti biodinamici, come i prodotti da agricoltura biologica che si trovano nella grande distribuzione, non hanno migliori caratteristiche nutrizionali, né hanno miglior cura dell'ambiente, prevedendo entrambi i disciplinari, biologico e biodinamico, ampie deroghe che consentono loro di utilizzare pesticidi di sintesi, che salvano le nostre colture dagli attacchi dei parassiti, consentendo a tutti di avere buoni e salutari

di interesse nazionale che vorrei tutelato da una politica basata sulle evidenze. Concludo senza nascondervi che da cittadina, prima ancora che da studiosa di scienze della vita, con esperienza ormai trentennale, provo sconcerto, sconforto e, quindi, dissento di fronte alla legittimazione per via parlamentare nell'ordinamento di uno dei Paesi più avanzati al mondo di pratiche antiscientifiche, esoteriche e stregonesche, specialmente se penso che, a sancire la superiorità del cornoletame sulle evidenze scientifiche, è la Camera alta del Paese che guida il G20, proprio nell'anno in cui per combattere la pandemia da Covid-19 il ruolo indispensabile della scienza è stato universalmente riconosciuto, celebrato e, anche in quest'Aula, osannato.

il verbo *colere*, che deriva dal latino, non significa solamente coltivare, ma anche abitare e venerare non certo i corni di vacca o le vesciche di cervo - ha ragione

quasi di una mistificazione. La narrazione dell'agricoltura è totalmente cambiata. Diecimila anni di storia sono stati messi in un cassetto e dell'agricoltura si è data una lettura bucolica (quasi fosse un retaggio del passato, una tradizione che non si rinnovava)

gli agricoltori e gli allevatori come se fossero la causa assoluta di tutti i mali dell'ambiente. In realtà, non è così e lo vedremo. Gli agricoltori in Italia rappresentano soprattutto esempi di sostenibilità

di terreni coltivati, la maggior parte è coltivata a foraggio o a pascoli, quindi non a produzioni antropiche importanti. Finiremo con il credere quello che un professor teorizza come la sindrome di Heidi, e cioè che l'agricoltura sia solamente le caprette che «ti fanno ciao» e non industrie e aziende agricole che negli anni hanno sviluppato una vera e propria capacità imprenditoriale che oggi le pone quale base di quel grande agroalimentare che fa della nostra Nazione una delle più importanti al mondo, se non la più importante. *(Applausi)*. Sono quasi 800 i nostri prodotti DOP e IGP riconosciuti universalmente in tutto il mondo, tanto che

di sola tradizione e che non si rinnova mai. Storicamente, in questa Nazione, specialmente nel secolo scorso, ma anche nell'Ottocento, quando nascevano le grandi case agroalimentari (la Buitoni, la De Cecco, la Barilla), tutte a cavallo tra il 1850 e il 1870, ma anche dopo, la politica agricola è stata oggetto di forte intervento pubblico. Come non citare Strampelli, il genetista agrario che rivoluzionò il frumento e portò le nostre produzioni per ettaro superiori a quelle di qualsiasi altro Paese nel mondo? Anche solo nel 1984, quando qualcuno prendeva in giro l'agricoltura attraverso i film - ne cito uno su tutti, «Il ragazzo di campagna» - in cui la campagna era descritta come qualcosa di antiquato, in quello stesso anno avevamo le rese per ettaro per il mais superiori a quelle degli Stati Uniti. Questo, però, non ce l'ha raccontato nessuno. Faceva comodo far credere che il *boom* industriale avesse convertito questa Nazione da povera e agricola in una industriale. E non è un caso che la maggior parte degli agglomerati urbani sia nata durante quel periodo, perché, finché davamo una lettura dell'agricoltura di abbiamo assecondato il depauperamento; abbiamo fatto sì che ci fosse quel travaso di forze e di capacità, anche intellettive e scientifiche, dalla campagna alla città. Nessuno può scordare il ruolo che hanno avuto negli anni agronomi agronomi come Draghetti, Gibertini o Edoardo Bassi, che batté le campagne a spiegare quali fossero le evoluzioni dell'agricoltura o la riforma agraria degli anni Cinquanta e Sessanta, con gli espropri, i fertilizzanti e i fitofarmaci, che dettero un impulso grandissimo

e, se la *farm to fork* dice che il 25 per cento delle superfici dev'essere dedicato all'agricoltura biologica, quel 75 per cento dovrà avere rese tali da consentirci non di fare la carne sintetico-scientifica, né di chiamare carne le polpette di soia, ma di avere una produzione tale da aumentare la nostra rendita per ettaro. Gli altri Paesi del mondo non stanno a dormire sull'agricoltura, fanno politica nazionale. Gli Stati Uniti hanno capito che il capito che il predominio dell'economia non esiste solo attraverso le armi, ma esiste anche attraverso la loro indipendenza alimentare. Lo sanno in Israele e perfino in Spagna; lo sanno in Cina, il cui *leader*, quando la la scure del Partito Comunista si abbatté sul padre, andò a lavorare in una fattoria, andò a lavorare in una fattoria, quindi conosce i problemi dell'agricoltura e sa anche che è soddisfacendo il fabbisogno alimentare che si rendono indipendenti i popoli. Lo sa la Russia, dopo che le abbiamo irrogato inique sanzioni, per cui si è strutturata per avere la propria indipendenza economica. In Italia, invece, abbiamo abbandonato tutto e lo abbiamo fatto anche a causa di qualche scandalo per il quale hanno pagato più gli agricoltori che i politici, e mi riferisco all'ammasso del grano.

un mazzo di catene che ci lega, ma è la bellezza da conservare. Conosciamo la tradizione, ma siamo sempre stati per un'innovazione che consenta di essere al passo coi tempi, com'è stato nei tanti periodi della politica agricola italiana, prima della guerra o nel dopoguerra, riportando al centro le istanze per la crescita e l'innovazione del Paese. Concentriamoci quindi sull'innovazione, sul recupero degli scarti, sulla depurazione delle acque contaminate, sui macchinari con sensori per rilevare le piante infestanti, sulle nanotecnologie, sulle serre automatizzate e su tutto ciò che ci riporta con i piedi ben ancorati alla tradizione, ma sicuramente

la grande distribuzione oggi paga un prezzo ed è su questo che dobbiamo lavorare all'interno della Camera alta, non su leggi che sono importanti, ma si traducono in un interesse per pochi. Dobbiamo garantire agli agricoltori un reddito equo che dia loro dignità,

In questo contesto, l'agricoltura biologica è l'unica via praticabile, se vogliamo davvero intraprendere la strada del *green deal* e del *farm to fork* europei, insomma se vogliamo davvero realizzare quella rivoluzione verde di cui tutti a parole ci facciamo promotori. Una reale transizione ecologica nello spirito europeo del *green deal* e del *recovery fund* passerà solo da una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari dei consumatori a favore di prodotti rispettosi dell'ambiente, della salute e del lavoro dell'uomo. Peraltro, l'agricoltura biologica ha un valore alto di mercato. Si consideri, infatti, l'incremento dei consumi registrato un anno fa, quando ebbe punte del 20 per cento in più a marzo-aprile, grazie proprio a una crescita nel valore tendenziale dello 0,2 per cento nel primo trimestre 2021. L'Italia vanta inoltre una delle maggiori quote nazionali di superficie agricola utilizzata nel biologico in Europa, con il 15,8 per cento, come hanno ribadito anche gli altri colleghi che mi hanno preceduto. Il nostro è il primo Paese in Europa e il secondo al mondo nell'esportazione di prodotti biologici, con oltre 2,6 miliardi di euro, circa il 6 per cento di tutto l'*export* agroalimentare nazionale. per potenziare questo settore non basta dichiararsi genericamente a favore del bio, ma bisogna essere concretamente accanto ai produttori biologici, garantendone la redditività e assicurando la più ampia partecipazione possibile a questo settore. Da qui è nata l'esigenza dei miei emendamenti, che poi illustrerò C'è però un altro punto che mi preme sottolineare, che nasce dall'esigenza di confutare le verità molto parziali diffuse in questi giorni sulla stampa dalla senatrice Elena Cattaneo, che mi ha preceduto, la quale ha presentato tre emendamenti per escludere dalla legge la parola «biodinamica», facendola passare per una cosa passatista e nemica dall'agricoltura, un ridicolo scientifico, come abbiamo sentito. Questo è assolutamente falso e, tra l'altro, penso che sia molto meglio il cornoletame del glifosato tanto caro alla senatrice Cattaneo, un contaminante estremamente nocivo di cui ella sembra farsi paladina, insieme al resto della chimica. Lo dimostra anche il fatto che lo scorso anno votò contro la mia mozione, approvata da tutta l'Assemblea, volta a escludere tale sostanza pericolosa dagli alimenti.

È importante far comprendere alla senatrice Cattaneo che, quanto alla definizione e all'uso dei preparati, vi sono regolamenti comunitari che riconoscono questi disciplinari proprio per una lunga tradizione di applicazione e che caratterizzano la gestione aziendale agroecologica a ciclo chiuso. Il richiamo necessario alla tradizione è coerente con la normativa UE (regolamento n. 848 del 2018), che in tema di biodinamica richiama proprio la tradizione.

Dalla prima regolamentazione dell'agricoltura biologica in Europa, avvenuta nel 1991, i regolamenti comunitari in materia di bioagricoltura includono sempre l'agricoltura biodinamica

Infine, il nuovo regolamento in materia di bioagricoltura (il n. 848, approvato il 30 maggio 2018) conferma la precedente giurisprudenza, ma inserisce l'agricoltura biodinamica nell'ambito di quella biologica,

È rilevante il riferimento alla tradizione: questo è un termine che ha una valenza peculiare in diritto e ha un pregio in chiave di diritto consuetudinario, proprio perché il legislatore ha inteso riconoscerlo. Non siamo di fronte a pratiche antiscientifiche, infatti la *review* delle pubblicazioni scientifiche sull'agricoltura biodinamica su riviste scientifiche soggette a referaggio, pubblicate per la Cambridge University Press nel 2009, evidenzia la consistenza della ricerca scientifica in agricoltura biodinamica, affermando che una buona parte dei risultati della ricerca dimostra gli effetti dei preparati sulla resa, sulla qualità del suolo e sulla biodiversità. La più recente *review* sul tema, nel 2018, ha esaminato 147 pubblicazioni su riviste scientifiche sottoposte a *peerreview* e ha evidenziato i risultati positivi emersi dall'analisi della letteratura. Il professor Pacini ha affermato che i sistemi biodinamici hanno dimostrato di avere il potenziale per essere superiori in date condizioni, sia quelli convenzionali, sia gli stessi biologici, per quanto riguarda la stabilità degli aggregati del suolo. Questi preparati, in determinate circostanze, hanno un impatto positivo sulla biodiversità. I sistemi biodinamici hanno un impatto positivo sull'utilizzo e sull'efficienza dell'energia, e allo stato dell'arte, nessuno è stato capace di rilevare quale principio scientifico sia alla base del funzionamento di questi preparati, né di dimostrare la loro supposta inconsistenza scientifica. Rudolf Steiner, che fu il fondatore dell'agricoltura biodinamica, studiò chimica presso il Politecnico di Vienna e conseguì il dottorato di ricerca in filosofia a indirizzo epistemologico, ebbe prestigiosi incarichi accademici, formulò una rigorosa teoria epistemologica, fu fondatore della corrente di pensiero denominata «scienza dello spirito» e fu uno dei padri della fenomenologia, insieme a Husserl, un suo collega di Vienna. A sviluppare sperimentalmente la biodinamica furono i più celebri scienziati, docenti universitari, allievi di Steiner. La prima formalizzazione matematica dei principi che sono alla base della biodinamica fu di un altro allievo di Steiner, il matematico George Adams, con laurea *ad honorem* in chimica a Cambridge. In quali istituti scientifici e università si ricerca e si insegna la biodinamica? Qualche esempio prestigioso: in Olanda l'Università di *Wageningen e* il Louis Bolk *Institut* sorto nel 1976 a *Driebergen;* in Germania, in tutte le facoltà di agraria viene introdotta la biodinamica e in particolare si insegna all'Università di Kassel,

Negli Stati Uniti, dal 2005 è stato costituito il **Biodynamic Research Network,** che federa diversi centri di ricerca operanti nella biodinamica in tutto il mondo. La biodinamica è quindi una pratica agricola non soggetta a restrizioni o brevetti e non consiste in una certificazione privata. La certificazione volontaria Demeter ha il fine di garantire in modo trasparente al consumatore l'applicazione del metodo agroecologico a ciclo chiuso. La Demeter in Italia è un'associazione non lucrativa di agricoltori italiani fondata nel 1984 per tutelare i frutti del lavoro agricolo e la trasparenza ai consumatori, fine nobile di un'agricoltura certificata. È una di quelle organizzazioni tipo che la dichiarazione ONU sui diritti degli agricoltori indica quale presidio per gli Stati che si impegnano a sostenere e a garantire i diritti contadini.

per ogni ettaro in agricoltura italiana coltivato in modo generale e convenzionale, c'è stato un reddito di 3.207; ogni ettaro coltivato ad agricoltura biodinamica ha prodotto un reddito per i nostri agricoltori di 13.309 euro. Il dato Il dato testimonia che le aziende biodinamiche sono indirizzate su colture di qualità, fortemente remunerative e pertanto costituiscono un modello con carattere di esemplarità di un'agricoltura italiana che vuol essere vocata alla qualità e all'alta e all'alta remunerazione per ettaro: altro che ridicolo scientifico! membri del Governo, colleghi, mi soffermerò solo su alcuni punti che ritengo peculiari della norma oggi in discussione. La norma recita che la produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale ed ambientale per lo sviluppo rurale, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e lo sviluppo sostenibile. Cari colleghi e Governo, grazie alla posizione e alla conformazione della nostra penisola con le sue isole, la varietà di climi, la diversità di altitudini e latitudini, la biodiversità in Italia esiste per natura. Quella biodiversità che va assolutamente tutelata e che occorre contrapporre all'appiattimento della più forsennata globalizzazione. *(Applausi).* Se aggiungiamo anche la nostra storia, la nostra grande cultura, unica al mondo in fatto di cibo e di cucina, il fatto che l'UNESCO abbia inserito la dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, definendola un insieme di competenze, conoscenze, riti, simboli e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, possiamo comprendere perché abbiamo il maggior numero di aziende di produzione e trasformazione con metodo biologico in Europa. Siamo fra i primi Paesi al mondo in termini di *export*, siamo fra i primi Paesi in Europa per superfici dedicate alla produzione biologica con circa due milioni di ettari, avuto negli ultimi anni i maggiori indici di crescita in Europa con i nostri agrumi, i nostri oli, i frumenti, i vini, gli ortaggi e quant'altro. Tutto ciò con un *e-commerce* in continua crescita, che facilita la diffusione dei prodotti anche delle più piccole aziende che creano tipicità, qualità e specialità. È infatti proprio su questa dimensione, sul parametro della botte piccola, che riusciamo a distinguerci trovando e creando mercato. In questo settore operano tante piccole e medie aziende, tante di quelle partite IVA presenti in tutti i settori dell'economia, sovente tartassate su tanti fronti che costituiscono il nerbo portante dell'economia italiana. Quelle aziende dove dipendenti, responsabile e titolare ogni mattina si devono armare di scudi, spade ed elmi per iniziare a combattere e ciò solo per produrre, creare e costruire in tutti i settori dell'economia italiana. Tornando però al tema dell'agroalimentare, mi vengono in mente, ad esempio, i *fancy food show*, dove gli *stand* dei produttori italiani sono sempre fra i più visitati e affollati. In questo contesto, ecco che prevedere il marchio del biologico italiano, che contraddistingue i prodotti ottenuti con metodo biologico con materie prime coltivate o allevate in Italia, diventa una garanzia in più per i consumatori e i produttori, soprattutto nell'ambito dell'*export*, dove tutti i prodotti del settore agroalimentare italiano, non solo quelli che seguono il metodo dell'agricoltura biologica, sono assai apprezzati - ahinoi - spesso in modo non lecito. Aggiungiamo anche che le normative, i regolamenti e i sistemi di controllo che abbiamo in Italia sono fra i più rigorosi al mondo e abbiamo il dovere di affermarlo e ribadirlo, anche contro un costume che ci vede spesso autocritici e finanche - mi sia consentito il termine crudo - autolesionisti. Questo disegno per rispondere anche a quello che ho sentito, stabilisce che ci possono essere anche altri metodi, che solo se rispettano quelli dell'agricoltura biologica possono essere dichiarati biologici. Poi, con una puntina di orgoglio, posso dire che il settore ha un grandissimo sviluppo nel Meridione d'Italia (quindi in Sicilia, in Calabria, in Campania e in Basilicata) e questo e questo - mi dispiace dirlo - va anche contro certe operazioni di qualche Ministero che ha tagliato i fondi verso il Sud. *(Applausi)*.

o allevate in Italia. 2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra stabiliti dall'Unione europea, contribuendo al raggiungimento dei propositi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il settore del biologico è in costante crescita e rappresenta una fetta importante del *made in Italy*, ponendoci tra i Paesi all'avanguardia in Europa. Le superfici agricole dedicate al biologico sono pari a due milioni di ettari, il 15 per cento della superficie agricola nazionale, localizzata soprattutto in Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia, con oltre 80.000 operatori impiegati nella filiera. Alla luce di questi numeri, lo Stato ha l'obbligo morale di promuovere e sostenere la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e piattaforme di aggregazione del prodotto e delle filiere. La recente emanazione del bando per la ricerca sul biologico, con uno stanziamento di 5 milioni di euro a partire da quest'anno e già previsto nella legge di bilancio del 2020, per la promozione del settore, dimostra quanto si stia puntando sulla sostenibilità ambientale dell'agricoltura. Tuttavia, non è ancora sufficiente e molto dev'essere ancora fatto. Tra gli obiettivi principali indicati dalla Commissione europea, vi sono il raggiungimento del 25 per cento delle superfici coltivate a metodo biologico e la riduzione di almeno il 50 per cento dei pesticidi: due assi strategici in cui l'Italia avrà un ruolo fondamentale. A nostro avviso, solo una visione agroecologica, ecosistemica e attenta alla qualità ambientale potrà ricreare un giusto rapporto tra uomo e ambiente. Auspico pertanto che le sensibilità presenti in quest'Aula possano contribuire, in un prossimo futuro, all'esito di un provvedimento legislativo più ampio sull'agroecologia, riconoscendo all'agricoltura il suo ruolo cruciale tra salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e qualità della vita. Lo sviluppo dell'agricoltura biologica assume grande rilevanza, tanto da rientrare tra gli obiettivi prioritari da perseguire, assieme alla riduzione della chimica utilizzata in agricoltura e nella zootecnia, al miglioramento del benessere animale e al contrasto della perdita di biodiversità. La realtà agricola organizzata secondo criteri di ecocompatibilità costituisce, dunque, il campo di indagine più appropriato per dare avvio a un rinnovamento culturale nella direzione dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, l'agricoltura biologica ha un ruolo rilevante. Secondo il Rodale Institute, tale metodo impiega il 45 per cento in meno di energia rispetto a quello convenzionale e fa un uso più efficiente dell'energia stessa, al contrario dei sistemi agricoli convenzionali, che producono il 40 per cento in più di gas serra. I suoli biologici, inoltre, hanno una funzione di *carbon sink*, che è mediamente quantificabile in mezza tonnellata per ettaro l'anno. In questo senso, l'agricoltura biologica offre agli agricoltori opzioni significative sia nelle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici sia in quelle di adattamento ai citati mutamenti. All'inizio del terzo millennio, dunque, ogni sforzo dev'essere dedicato a riorientare il comune patrimonio di conoscenze nella direzione di un umanesimo agroecologico ed ecocompatibile. Per incrementare questa tendenza, occorre organizzare al meglio i distretti biologici e la filiera produttiva, con un supporto sia tecnico sia commerciale. Bisogna puntare sulla transizione digitale, utilizzando ad esempio la tecnologia *blockchain* per tracciare i prodotti agroalimentari. I dati elaborati dal Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB) lo dimostrano: dal 2010 gli ettari destinati alle colture biologiche sono aumentati di oltre il 75 per cento e il numero degli operatori del settore di oltre il 65, mentre i consumi di prodotti bio sono più che raddoppiati dal 2013 ad oggi. Si tenga presente che il biologico è il solo metodo agricolo chiaramente regolato e riconoscibile agli occhi dei consumatori grazie alla sua certificazione, che è stata fondamentale per l'espansione del mercato, dando un'identità a quei prodotti. A tal riguardo, tra le novità più interessanti contenute nel disegno di legge in discussione vi è la creazione di un marchio bioitaliano, che garantirà ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che provengono dalle filiere biologiche completamente italiane. Sono previsti anche piani di azione per il settore e per le sementi, un fondo di sostegno alla ricerca, alla formazione e alla promozione di accordi quadro e alle intese di filiera. I cibi biologici prodotti senza l'impiego della chimica sono più sani e garantiscono *standard* di salute più elevati. Lo ha affermato con chiarezza il commissario europeo all'agricoltura Janusz Wojciechowski durante la presentazione del Piano d'azione biologica dell'Unione europea, aggiungendo che, nella sua visione ideale, tutta l'agricoltura europea dovrebbe essere bio. Concludendo, l'agricoltura biologica ha un impatto ambientale inferiore rispetto alla produzione convenzionale e c'è una crescente domanda di cibo biologico, sia per l'Europa sia a livello globale, poiché sempre più persone cercano cibo sano. A conferma di quanto detto, nei giorni scorsi è stato presentato dalla Commissione europea il nuovo Piano d'azione 2021-2027 per la transizione agroecologica dell'agricoltura europea. Gli obiettivi sono individuati dal *green deal*, dalle strategie comunitarie *farm to fork* e a difesa della biodiversità: triplicare le superfici agricole coltivate a biologico e dimezzare l'uso di pesticidi e antibiotici Il Piano sostiene i consumi, puntando a una maggiore diffusione dei prodotti biologici nelle mense pubbliche e scolastiche. Al tempo stesso, il miglioramento della tracciabilità dei prodotti biologici contribuirà a prevenire le frodi e aumentare la fiducia dei consumatori. Sul fronte della produzione, è necessario incentivare gli agricoltori al passaggio dal convenzionale al biologico, attraverso azioni di sostegno. Attualmente, infatti, solo l'1,8 per cento (pari a 7,5 miliardi di euro) della politica agricola comune è utilizzato per l'agricoltura biologica, mentre per la sostenibilità del settore i distretti bio potrebbero unire il tema dell'agricoltura a quello del turismo e della valorizzazione territoriale. L'Italia su questi fronti può giocare un ruolo da protagonista. Su questo percorso dobbiamo quindi continuare a lavorare per andare in questa direzione. Infine, voglio citare le parole dell'ex *premier* Giuseppe Conte, che nel giorno del voto di fiducia al suo secondo Governo, oltre a considerare centrale e decisivo il comparto agricolo, si è espresso con favore nei confronti dell'approccio biologico in un passaggio del suo discorso, affermando: «È necessario sviluppare la filiera agricola biologica, le migliori pratiche agronomiche, accrescere la qualità del territorio, sostenere le aziende, investire nella ricerca sulle coltivazioni, con particolare attenzione all'uso efficiente della risorsa idrica». Colleghi, oggi è un giorno che, inevitabilmente, potrà restare nella storia del nostro Paese quale punto di svolta verso un futuro nettamente diverso e distinto dalle abitudini nocive del passato, secondo quella svolta verde, amica dell'ambiente, che ci chiedono da tempo i giovani del movimento che garantisca a tutti noi di vivere in un pianeta più sano ed equilibrato, scevro da pratiche intensive e inquinanti. Con questo provvedimento legislativo l'Italia potrà rivestire un ruolo da protagonista in Europa, rafforzando la *leadership* di produttore nel settore agroalimentare e, e, in particolare, in quello biologico. Questo disegno di legge rappresenta un nuovo modo di approcciarsi alle prossime sfide globali, in cui pensiero e azione sono conformi al paradigma ecologico.

di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica». Quindi tutti coloro che rispettano l'agricoltura biologica sono equiparati. Abbiamo scritto anche: «Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo».

permacultura ed altri sistemi stanno andando in questa direzione; quando avranno maturato tale convinzione e faranno richiesta al Ministero, riceveranno lo stesso identico trattamento previsto per l'agricoltura biologica. Di questo stiamo parlando, non di altre questioni. Per quel che ci riguarda, a noi interessa che gli alimenti che vengono prodotti per i nostri consumatori rientrino nel pieno rispetto delle regole previste per la salute e la salubrità dei prodotti e nel rispetto di tutti i regolamenti previsti. Dopodiché, se qualcuno vuole farlo con le lune che ritiene o convinto che ci siamo preparati che aiutano, purché non siano tossici, a noi non crea nessun problema. Perché dobbiamo azzoppare un sistema che vale centinaia di milioni di euro, esporta il 95 per cento del prodotto e garantisce agli agricoltori un reddito di 13.000 euro ad ettaro? Credo sia

quale stanno credendo e investendo moltissime aziende agricole. Non costringiamo nessuno a fare nulla, ma riteniamo che, se qualcuno opta per questa soluzione, debba avere il rispetto e la dignità che questo tipo di agricoltura merita,

non dobbiamo fingere che su questi temi l'agricoltura e l'Unione europea abbiano preso un abbaglio. La scelta che l'Unione europea ha fatto è di grande buon senso, molto rispettosa della qualità dei nostri suoli e della nostra agricoltura, e credo che abbia fatto bene a intraprendere questo tipo di strada. È legittimo che qualcuno la pensi in modo radicalmente diverso; non voglio né convertire né convincere nessuno. Credo però che abbia piena dignità in questa stagione e in questo Paese l'approvazione di una legge sull'agricoltura biologica, perché - lo ripeto - si tratta di un fenomeno crescente e migliaia di aziende legano a questa tipologia di agricoltura

innanzitutto per ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti e i membri della Commissione agricoltura che hanno lavorato al testo, ai fini della sua approvazione. Mi preme sottolineare che questo è un settore in cui l'Italia è prima in Europa non soltanto per la produzione, ma anche per la superficie dedicata (16

condivido il 99 per cento degli interventi che sono stati fatti, perché poi tutti si sono pronunciati a favore del disegno di legge, e questo è un dato importante.

le aziende biodinamiche attualmente in Italia sono 4.500 e rappresentano una realtà importante, della quale l'agricoltura in generale deve tener conto.

l'emendamento 1.200 elimina dal comma 3 dell'articolo 1 il riferimento specifico all'agricoltura biodinamica che trovate nel testo, poiché si tratta di una pratica priva di riferimenti scientifici, fondata su principi esoterici e stregoneschi. In ogni caso, poiché, come è specificato nello stesso comma 3, esiste una procedura di equiparazione fissata dal Ministero delle politiche agricole, cui ogni metodo rispettoso dei disciplinari biologici può provvedere a conformarsi, è irragionevole citare esplicitamente solo quello specifico tipo di agricoltura, come possibile sottoinsieme di metodi equiparabili al bio. Ritengo che questo regime di eccezione e di tassonomia esplicita per la sola biodinamica sia biodinamica sia un elemento di confusione per il cittadino consumatore e anche una discriminazione verso le altre pratiche agricole, comunque rispettose già oggi dei disciplinari del biologico, che non godranno di esplicito riconoscimento, e che segnali anche un evidente *bias* cognitivo cioè un malcelato favore preconcetto verso la pratica esoterica del biodinamico. Come vedremo, questo preconcetto trova compiuta esplicitazione all'articolo 5, che prevede che solo il sottoinsieme della pratica biodinamica abbia diritto ad una rappresentanza specifica di propri portatori di interesse al tavolo tecnico per la produzione biologica. Per questi motivi, colleghi, vi chiedo di valutare attentamente l'emendamento e di considerare di votare in suo favore. Infine, voglio ribadire che, se questo emendamento fosse approvato, non vi sarebbe assolutamente nessuna conseguenza per i coltivatori biodinamici che rispettino i limiti e le regole del biologico e il legislatore si risparmierebbe di dare dignità di legge a idee che, per quanto suggestive, si rapportano alla realtà delle cose tanto quanto possono farlo gli oroscopi.

Signor Presidente, l'agricoltura biologica è una grande opportunità per il nostro Paese e, con il disegno di legge in esame si stabiliscono regole certe, a tutela della salute dei cittadini e dei prodotti.

tutto diversa è invece l'agricoltura biodinamica, che è un insieme di pratiche pseudo-scientifiche, basate sulla visione spirituale del mondo, elaborata dal teosofo ed esoterista Rudolf Steiner, nato nel 1861. Vorrei correggere il collega senatore intervenuto in precedenza: Rudolf Steiner non si è mai laureato in chimica o in ingegneria, ha frequentato qualche corso all'Università di Vienna e poi si è laureato in filosofia. Gli studi scientifici effettuati non hanno rilevato incremento di qualità tra i prodotti biodinamici e quelli coltivati con i consueti metodi biologici. In compenso, una camomilla preparata mettendola all'interno dell'intestino di bue sotterrata per qualche mese potrebbe poi diventare, sul tavolo del consumatore, una bomba, ad esempio a causa dell'escherichia coli. Questo professore ha fatto otto lezioni lezioni sull'agricoltura nel 1925; da qui è nata questa teoria biodinamica. Io sono molto aperta a qualsiasi teoria innovativa; questa non è innovativa, ma comunque è saltata fuori, forse perché questo metodo olistico fa molto piacere al giorno d'oggi a qualcuno. Nel pieno rispetto di tutte le 4.000 aziende che hanno prodotti biodinamici, penso che esse meriterebbero un occhio di riguardo a sé

questo importante e atteso provvedimento, che non prevede solo la produzione agricola e agroalimentare, ma anche l'acquacoltura biologica, con tutto quello che ne deriva. Vorrei ringraziare il senatore Mollame per l'egregio lavoro svolto in Commissione e per il lavoro e la discussione che sono stati fatti in merito a questo provvedimento sia in Commissione che anche al Ministero. In merito proprio a questo emendamento, mi preme precisare con fermezza che la questione del metodo biodinamico da inserire in questo provvedimento ha visto una grande discussione in Commissione, perché tutti gli interrogativi posti dalla collega Cattaneo sono stati abbondantemente affrontati. Noi abbiamo risolto il problema inserendo in seconda lettura, presso la Commissione

dell'agricoltura biologica sono equiparati. L'equiparazione non è pertanto automatica, ma è sottoposta alla richiesta dell'interessato, previo il rispetto del metodo biologico così come previsto dalle norme europee e dalla norma nazionale. Naturalmente c'è la discrasia della rappresentanza ai tavoli. Ma, nel momento in cui qualsiasi metodo che viene utilizzato per produrre del cibo rispetta il disciplinare del biologico nazionale, perde la sua prima caratteristica (che potrebbe essere biodinamico o qualsiasi altra forma) e diventa a tutti gli effetti biologico, sia per il regolamento europeo che per il regolamento nazionale. Ecco perché io dico che, rispettando tutte le eccezioni sollevate dalla senatrice Cattaneo, questi interrogativi sono stati già risolti con l'aggiunta che la Commissione agricoltura del Senato ha fatto al testo che ci è arrivato dalla Camera.

Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sugli emendamenti. Inizio dicendo che Fratelli d'Italia fin dall'inizio, all'interno

provvedimento rispetto al testo uscito dalla Camera. Sicuramente abbiamo fatto un buon lavoro. Nello specifico, noi di Fratelli d'Italia avevamo già la questione dell'equiparazione fra il biologico e il biodinamico. Infatti avevamo presentato l'emendamento 1.10, con il quale chiedevamo addirittura la soppressione del comma 3, che equipara l'agricoltura biologica all'agricoltura biodinamica. Ora, non entro nel merito delle varie pratiche e dei principi; il nostro è un ragionamento puramente legislativo e tecnico. Infatti qui si indicava in maniera generica il rispetto delle disposizioni del regolamento UE in materia di agricoltura biologica, senza definire il metodo dell'agricoltura biodinamica, limitandosi a prevedere solo l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari. In assenza pertanto di specifiche indicazioni normative nell'articolo 1 del disegno di legge si proponeva, con il nostro emendamento, la soppressione del comma, in quanto l'agricoltura biodinamica è frutto solamente di autoregolamentazione privata e non risponde a regolamentazioni normative europee, né nazionali. l'agricoltura biologica è regolata dai regolamenti europei n. 834 del 2007 e n. 848 del 2018, mentre non sussistono disposizioni legislative con le quali poter procedere a un'equiparazione. Per questi motivi,

Ciò che mi sorprende è la caparbietà con cui si è voluto introdurre l'agricoltura biodinamica nel disegno di legge in esame. Il mio sospetto è che avere tanti enti regolatori, incluso quello del biodinamico, possa far comodo a molte associazioni di categoria. Non vi è alcun motivo per introdurre il termine biodinamico in un disegno di legge sull'agricoltura biologica. Con il massimo rispetto per tutte le discipline spirituali che caratterizzano il mondo agricolo (ci sono non solo la biodinamica, ma tante altre

Signor Presidente, l'emendamento 5.100 da me presentato è finalizzato a ripristinare il numero dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, che oggi nel comitato sono cinque, mentre il comma che andiamo a emendare ne prevede quattro. Così come congegnato, se approviamo il testo in questo modo, il provvedimento affiderà nelle mani di un solo soggetto la gestione vera e propria dell'intero comparto biologico. È per questo che in Commissione avevo presentato due emendamenti utili a rendere più democratico il provvedimento. Gli emendamenti, ammessi in Commissione bilancio, sono decaduti poi in Commissione agricoltura, in considerazione del parere contrario del Governo e del relatore. L'importanza che assumerà questo comparto nei prossimi anni e l'imponente massa di finanziamenti che sarà destinata al settore ci fa ritenere che la platea da coinvolgere debba essere la più vasta possibile e che vada raggiunto il coinvolgimento del maggior numero di strutture operanti da anni nel settore. Dobbiamo, quindi, puntare a rendere più democratica la gestione economica di questo comparto, che oggi assume un'importanza strategica per le prossime scelte anche a livello comunitario. Secondo la visione riportata nel testo, non è pensabile che la platea da coinvolgere nel tavolo tecnico presso il Ministero debba essere ridotta rispetto a quella che è già attualmente prevista nel tavolo compartecipato.

Presidente, l'emendamento 5.200, come ho anticipato poc'anzi, mira a rimuovere dall'articolo 5 il riferimento specifico alla presenza nel tavolo tecnico di un portatore di interesse del cosiddetto metodo biodinamico. Faccio questo per due motivi. Di fatto, tutti i metodi equiparati all'agricoltura biologica, in quanto a essa equiparati, come da articolo 1, trovano già i propri rappresentanti nei membri che partecipano al tavolo per conto delle associazioni maggiormente rappresentative della produzione biologica. citare esplicitamente la presenza di un rappresentante del metodo biodinamico significa privilegiare nella rappresentanza i portatori di interesse di tale agricoltura esoterica rispetto a quelli degli altri metodi equiparabili al biologico. La previsione di una rappresentanza esclusiva dedicata a una sola delle possibili sottocategorie della coltivazione biologica, cioè la biodinamica, crea davvero una discriminazione rispetto ad altri metodi. Discriminazione, peraltro, fatta fatta per legge, quindi destinata a durare nel tempo, che, per essere superata, necessiterebbe di un altro intervento legislativo volto a eliminare la disparità o a riservare ulteriori scranni alle nuove sottocategorie del biologico. Chiedo quindi come sia possibile che questo sia il tipo di rappresentazione degli interessi del settore che davvero ritenete che debba esser presente al tavolo tecnico istituito da questo articolo. Per queste ragioni

solo ed esclusivamente come un qualcosa di particolare. A me sembra che invece ci sia un atteggiamento esoterico contro la biodinamica: chi vuole fare qualcosa all'interno della propria azienda lo può fare a prescindere e lo potrà fare anche

tocca un tema particolarmente importante, anche in questa terza fase della legislatura: quello della transizione ecologica. Abbiamo un super Ministero che si impegna a lavorare sulla transizione ecologica, ossia per una modernizzazione dei metodi e per una visione e una valutazione scientifica del fondamento delle decisioni che si prendono. Non a caso, nel tavolo tecnico che viene istituito con questo articolo, ci sono

molto succosa, se volete, per fare dell'ironia su ciò che è stato, ma che comunque appartiene a un passato culturale, quando le metodologie erano puramente improvvisate, quando ci si disponeva ad affrontare un problema senza averne la soluzione, ma senza averne nemmeno capito l'esatta natura, per cui qualunque cosa poteva essere fatta, perché qualunque cosa forse avrebbe potuto intercettare o il consenso degli Dei o quello delle stelle. A me sembra che mescolare, in un tavolo che vuole davvero guardare alla modernizzazione dei processi, persone che sono portatrici di interessi di categoria, ma anche di microcategoria, ma soprattutto soprattutto di una cultura che stiamo in qualche modo cercando di superare per andare oltre proprio con la transizione ecologica, mi sembra francamente un po' ridicolo. Pertanto io voterò in dissenso dal Gruppo e a favore dell'emendamento 5.200 della collega Cattaneo.

Ci sono tanti modi di fare agricoltura; gli agricoltori italiani la fanno in tanti modi cercando di ridurre i pesticidi; alcuni guardano la luna, mio suocero guardava le fasi lunari, io stessa mi impegno in agricoltura e faccio delle pratiche che sono anche propiziatorie. Tuttavia, inserirle in un disegno di legge è veramente inopportuno e lo si fa perché questo è un disegno di legge lobbistico, dove l'estrema destra si connette esotericamente con il *radical chic* dell'esoterismo e della della spiritualità agricola, in cui nessuno sa cosa significa vivere di agricoltura. Io lo so perché vengo da una famiglia che è vissuta di agricoltura e non posso tollerare che si facciano queste stranezze stranezze nei disegni di legge che devono sostenere l'agricoltura in un periodo difficilissimo e lo devono fare rispettando l'ambiente, riducendo al minimo l'uso dei pesticidi, ma non cedendo alle *lobby* di tutti i generi che piacciono tanto a quest'Assemblea.

si restringono i portatori di interesse che si occuperanno di un settore innovativo che dovrebbe essere aperto a tutti e non solo a quattro soggetti.

questo emendamento all'articolo 8, che tratta del Piano nazionale delle sementi biologiche, mira ad eliminare la parola «biodinamica» alla fine del primo comma e la ragione è evidente: si tratta di una specifica non necessaria, essendo di per sé evidente che se la biodinamica è equiparata al biologico, essendone una sorta di sottocategoria con aggiunte esoteriche e stregonesche, beneficerà comunque della disciplina di questo articolo dedicato al Piano nazionale delle sementi biologiche. Ancora una volta, il riconoscimento espresso è una operazione di *marketing* del *brand* biodinamico e delle sue attività inserito in un contesto legislativo a cui confido questa Assemblea non voglia prestarsi. Chiedo quindi che voi consideriate con favore questo emendamento e siccome questo è l'ultimo emendamento dei tre che ho presentato, tutti volti alla stessa finalità, vorrei aggiungere qualche riflessione. La finalità dei tre emendamenti è risparmiare a questa Camera la responsabilità di inquinare l'ordinamento italiano con qualcosa che con le prove, la realtà e la scienza non ha nulla a che fare, tra l'altro in un settore importantissimo; evitare a questa Camera di fare lo stesso errore commesso nella conversione del decreto della sperimentazione su Stamina e cioè aprire a una forma di legittimazione di attività esoteriche esoteriche e stregonesche che lucrano sull'ignoranza dei consumatori. Tenete conto, poi, che tali organizzazioni da domani potranno farsi forte della *Gazzetta Ufficiale* per rivendicare una loro solidità.

esattamente la confusione che si creò con Stamina e voi tutti - perché alcuni di voi c'erano - conoscete la fatica e il dolore che costò smascherare Stamina,

una truffa fondata sulla credulità popolare, alimentata dai *media*, avallata da alcuni tribunali del Paese, a cui il Parlamento aveva risposto supinamente, aggravando quel che invece andava fermato.

sviata dalla discussione in Aula e fu proprio questa Assemblea poi a porre rimedio. Costò mesi e un'indagine conoscitiva voluta dalla collega precocemente scomparsa senatrice Emilia De Biasi, disse, terminata all'indagine conoscitiva, alla conferenza stampa, senza mezzi termini, che il Parlamento aveva sbagliato. Spererei che non si voglia sbagliare ancora così platealmente. Nella vicenda Stamina la Camera, grazie all'attivismo di alcuni, limitando i danni potenzialmente in grado di far saltare il Servizio sanitario nazionale, corresse quanto approvato dal Senato. Confido che la dinamica virtuosa del bicameralismo si ripeta anche per questo disegno di legge. Concludo ponendovi qui in Aula, pubblicamente, la domanda che decine di eminenti studiosi e imprenditori contrari a questa legge hanno posto in una lettera inviata ieri a tutti i senatori. È una domanda essenziale per decidere dei temi in discussione, che potrà orientarci nel voto di quest'ultimo emendamento. La domanda è se può il Paese di Galileo Galilei sostenere economicamente, con denaro pubblico, pratiche magiche, peraltro facenti capo ad un marchio registrato estero. Personalmente, tra Galileo Galilei e i novelli alchimisti, ho ben chiaro chi e cosa sostenere nell'interesse dei cittadini: il metodo scientifico. Spero che in queste settimane, in cui grazie alle vaccinazioni il Paese comincia a rivedere la luce dopo più di un anno di buio, la risposta possa essere chiara e univoca anche per ciascuno di voi.

che a parte l'agricoltura biodinamica, esistono tante agricolture. Esiste la sinergica che è scientificamente comprovata e non usa pesticidi perché usa una combinazione di piante che si autotutelano a vicenda. Esiste la permacultura. Esistono delle sperimentazioni sul nostro territorio che sono splendide, non usano pesticidi e non sono citate nella legge al nostro esame. Ricordo a chi si proclama vegano, vegetariano e *no* *animal* che questa è l'unica forma di agricoltura che prevede che per fecondare la terra serva uccidere una vacca vergine. Questo vorrei ricordare. Allora chi mangerà vegano biodinamico sappia che comunque ha ucciso una vacca, giusto per smascherare l'ipocrisia di chi vede in questa roba esoterica la soluzione per i mali del mondo. Non lo sono, esistono pratiche molto più scientifiche, molto più legittime e molto più importanti - che dovevano essere citate nella legge io ho cercato di proporre - che sono appannaggio dei giovani, dei ragazzi, senza marchio registrato, a differenza di questa che è un marchio tedesco e che invece non sono state prese in considerazione. Voterò a favore dell'emendamento 8.200 perché l'Assemblea sta facendo di nuovo un errore, come nell'epoca Stamina;

perché mi sembra che equiparare l'agricoltura biologica, dietro la quale ci sono ricerca, innovazione, formazione e tecnologie, all'agricoltura biodinamica, significhi veramente svilire l'importanza dell'agricoltura biologica e delle possibilità di sviluppo nel nostro Paese.

ciò mi preoccupa molto. Propongo pertanto di riportare il testo in Commissione, fare le audizioni dovute, con le associazioni e i comitati scientifici, e poi riportare il disegno di legge in Assemblea.

un'altra percentuale, quella dei terreni tradizionali o dei terreni industriali, su cui si potrà lavorare con l'innovazione, con le tecnologie e la tecnica a disposizione in questo millennio per riuscire ad aumentare la redditività e la produttività, soprattutto dei nostri terreni. Come dobbiamo fare? Dobbiamo farlo con quel concetto di sostenibilità che oggi

Gli agricoltori italiani, nonostante uno Stato cieco e quest'Aula spesso sorda, sono avanti anni luce rispetto a quello che delibera l'Europa. Quindi, cerchiamo non dico di sostenerli, perché mi sembra evidente il disinteresse con il quale si trattano temi come quelli in esame, ma almeno di non ostacolarli,

è una pratica di nicchia, una pratica importante. Non è tutta l'agricoltura, ma è una delle tante agricolture che fanno grande questa Nazione, ma che non hanno nulla a che vedere con pratiche e riti come quello delle corna delle vacche o delle vesciche dei cervi, che invece l'agricoltura biodinamica purtroppo introduce.

Presidente, nella confusione dell'Aula, si sente davvero male e quindi abbiamo commesso questo errore. PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. È il motivo per cui delle volte cerco di non andare velocissima, per dare a tutti la possibilità di comprendere.

Molti hanno posto il tema del perché l'agricoltura biologica sia presente nei vari tavoli. Ad oggi l'unica forma di agricoltura formalmente e giuridicamente equiparata a quella biologica è quella biodinamica.

l'emendamento è finalizzato al riconoscimento di più organizzazioni professionali, laddove nel testo del provvedimento viene riconosciuta, di fatto, una sola organizzazione, e sappiamo tutti qual è. Chiedo, quindi, vivamente all'Aula di votare a favore della democrazia economica e della partecipazione. Quanto previsto all'articolo 14 è un modo inconcepibile di concentrare tutto il *business* nelle mani di un solo soggetto, creando un vero e proprio gruppo di potere cui verrebbe consegnato l'intero settore nei prossimi anni. La preoccupazione, pressoché certezza, è che si possa arrivare a una politica di monopolio, considerando le percentuali del 30 per cento richieste; percentuali che sembrano favorire un solo gruppo a scapito di quell'universo, cioè del 70 per cento rimanente, che resterebbe fuori, ma pesantemente condizionato dall'unico soggetto riconoscibile per legge dal Ministero, che tutti conoscono. Così come scritto, l'articolo 14 avrebbe ripercussioni anche sui biodistretti che abbiamo approvato nell'articolo 13. Invito, quindi, vivamente l'Aula a riconoscere il valore e la funzione della democrazia nel nostro Paese e ad approvare questo emendamento.

e, attraverso un progetto di economia circolare, dagli scarti recupera una pasta che può essere utilizzata sia in pasticceria che nella cosmesi per le creme di bellezza. Elisabetta invece, dopo la laurea in tecnologie alimentari, produce confetture e succhi biologici con la frutta che lei stessa coltiva, attraverso un metodo sostenibile senza anticrittogamici. sono solo alcune delle storie di tanti giovani produttori che in modo pionieristico hanno deciso di scegliere un tipo di coltivazione con minor impatto sull'ambiente e sulla salute. Con il disegno di legge che stiamo per votare, diamo alcune certezze e una cornice legislativa di riferimento ai tanti agricoltori che, come Elisabetta e Lorenzo, hanno avuto il coraggio e l'intraprendenza di dedicarsi con metodo biologico alla produzione agricola, agroalimentare o all'acquacoltura. in esame, scritto a più mani dalla collega Maria Chiara Gadda con alcune associazioni di categoria e con la filiera agroalimentare, il Parlamento offre uno strumento utile a un settore che si ritrova a essere centrale in una fase di particolare attenzione per l'ambiente e l'ecologia. Quello della produzione biologica è un comparto importante e competitivo, che è stato anche più capace, rispetto ad altri settori, di resistere alla crisi di questi anni; è un comparto che ha ancora grandi potenzialità e che attende da anni una normativa compiuta. Nel testo la produzione biologica viene riconosciuta come attività di interesse nazionale, con una funzione sociale e ambientale. La produzione biologica viene definita come un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e la salvaguardia delle risorse naturali. Grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti e alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, come pure alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Credo che non sia utile scatenare battaglie ideologiche tra produzioni con metodo biologico e convenzionale, perché oggi per tutti l'obiettivo è ridurre l'impatto della chimica nel suolo. Quello del biologico è un comparto regolamentato anche a livello di Unione europea, e per l'Italia rappresenta un settore importante in termini di PIL, di occupazione e di *export*. Il disegno di legge, insieme al Piano strategico e a un adeguato sistema di controlli, serve a rendere più strutturato un settore che può crescere ulteriormente perché, tra l'altro, intercetta anche i bisogni di acquisto e di consumo dei cittadini. Il biologico italiano ha inoltre una storia di successo e lo dicono i numeri anche in termini di fatturato. L'Italia è uno dei principali produttori europei di questo tipo di coltivazione. Secondo le ultime stime, sono oltre 76.000 le aziende del comparto biologico nel nostro Paese; coltivano attorno ai due milioni di ettari, con un fatturato di circa 3,5 miliardi di euro l'anno. Pertanto, il bio non è più settore di nicchia, ma è sempre più spesso il frutto delle scelte di impresa che rappresentano una quota rilevante del *made in Italy*. Con questo provvedimento si istituisce anche un marchio biologico italiano che valorizza le coltivazioni agricole del nostro Paese, rendendo riconoscibile ai consumatori l'origine della materia prima agricola. Viene inoltre fornita una regolamentazione ai distretti biologici, che possono rivelarsi uno strumento utile nell'ottica delle politiche del territorio, affinché non vi siano solo i singoli agricoltori, ma si possano anche costruire dei distretti con il compito di adottare politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente e di conservazione del suolo agricolo. Questa regolamentazione potrà incidere positivamente sui territori creando dei cicli virtuosi che possono coinvolgere anche il settore enogastronomico. Le aziende agricole biologiche in Italia sono localizzate principalmente in aree collinari e montane, soprattutto in Sicilia, Calabria, Puglia. Da analisi recenti dei dati, emerge che spesso l'attività da agricoltura biologica si accompagna a un ritorno dei giovani all'imprenditoria giovanile proprio in quelle zone; il che può essere strategico in una fase in cui puntare sui giovani può aiutare a risollevarci da un'emergenza pandemica che ha messo in ginocchio moltissime attività, proprio e soprattutto anche in aree limitrofe come quelle. Intanto, il consumo di prodotti biologici, da alcuni anni a questa parte, sta riscontrando una crescita costante, che prende sempre più piede anche nella grande distribuzione con ottimi risultati. Molti consumatori sempre più spesso fanno attenzione alla qualità dell'alimentazione, privilegiando l'acquisto di prodotti meno trattati chimicamente e quindi più sani. Si tratta di una tendenza che è aumentata, tra l'altro, anche durante la pandemia da Covid-19. Dietro a ogni singolo frutto che mangiamo, dietro a ogni verdura e a ogni pietanza, c'è un mondo, una filiera di passaggi, di persone e di aziende. Credo che ciò sia una grande sfida per la nostra agricoltura nel suo complesso e, al suo interno, proprio per l'agricoltura biologica. La consapevolezza di un numero crescente di consumatori finali di volersi nutrire con prodotti di qualità, salubri e ottenuti con modalità sostenibili, è un grande valore aggiunto per la qualità dei prodotti e per la tutela dei terreni e dell'ambiente. Questa consapevolezza e la conseguente richiesta possono rivelarsi uno straordinario volano di sostegno economico proprio per le terre agricole con maggiori difficoltà. Credo che questa sia una bella pagina dell'attività legislativa nei confronti dei tanti coltivatori che, come Elisabetta e Lorenzo, scelgono la strada dell'agricoltura biologica con coraggio e dedizione e anche nei confronti di quei consumatori che decidono di prestare maggiore attenzione a ciò che consumano. Verso queste persone e verso quegli imprenditori abbiamo il dovere oggi di approvare il decreto-legge

doveva essere in un primo momento discusso, emendato e poi approvato, prima in sede redigente, poi in sede deliberante e infine, per procedure di natura tecnica, praticamente a lavoro concluso, è stato rimandato ancora in Commissione, in sede referente, per venire finalmente in Assemblea per il voto finale. Niente di male, anzi penso che il disegno di legge in esame, per l'importanza del tema, aveva ed ha il diritto e la dignità di essere discusso e approvato in Il secondo motivo che mi ha portato ad usare il termine "finalmente" è legato a un tema più generale: finalmente discutiamo di nuovo di un provvedimento di iniziativa parlamentare. Finalmente - lo ripeto - ridiamo il giusto significato al ruolo del Parlamento: dopo mesi di decreti governativi, torniamo, almeno oggi, a discutere un disegno di legge di iniziativa parlamentare. Onorevoli colleghi, quella che dico non è una banalità, ma è semplicemente quanto tutti i Gruppi parlamentari hanno detto, di certo in momenti e con ruoli diversi dal presente, lamentandosi del fatto che il Parlamento è stato scippato dalle sue prerogative, diventando solo un passacarte del Governo di turno. Allo stesso modo tutti hanno detto - e tutti se ne sono lamentati che di fatto è stato abolito il bicameralismo perfetto, riducendo il lavoro di una delle due Camere a semplice attività di ratifica di quanto fatto dall'altra. Tutti lo hanno detto, ma Fratelli d'Italia è l'unico partito che lo ha sempre detto e che può dirlo anche oggi con la stessa coerenza di ieri.

Il settore del biologico del nostro Paese ha registrato, negli ultimi anni, una crescita esponenziale, come confermato dai dati diffusi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Infatti, dal 2010 ad oggi, sono oltre 800.000 gli ettari che in Italia sono stati convertiti al biologico, con una crescita percentuale, negli ultimi anni, di oltre il 70 per cento. Si tratta comunque di un dato che, già da solo, rende perfettamente l'idea di come si stia orientando il mercato, che deve spingerci tutti ad un'attenta analisi e all'adozione di misure adeguate, per stare al passo con la spinta impressa a questo settore. Il biologico in Italia viene coltivato su un numero importante di ettari da oltre 75.000 imprese. L'Italia conferma di essere quindi uno dei principali Paesi in Europa per questo tipo di coltivazione. Anche i dati sui consumi di biologico in Italia segnalano importanti indici di crescita, con un incremento generalizzato per tutte le referenze biologiche vendute sia nella grande distribuzione, sia nei negozi specializzati. L'Italia è inoltre ai primi posti in Europa per l'*export* di prodotti di origine biologica e - secondo una ricerca condotta dall'ISPRA - il fatturato oltre frontiera è superiore a un miliardo di euro, un importo che rappresenta più di un terzo del giro d'affari complessivo del biologico italiano. Proprio per queste ragioni ritengo, e tutti noi di Fratelli d'Italia riteniamo, che il provvedimento oggi in esame sia di estrema importanza, anche in base ai numeri che ho appena elencato, in quanto ha la funzione di disciplinare un settore in forte espansione, quale è appunto quello dell'agricoltura biologica. Il provvedimento ha l'obiettivo - come si dice anche nel testo - di favorire e promuovere iniziative volte all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione delle filiere e dei prodotti biologici, perfettamente in linea con gli obiettivi europei per la realizzazione del PNRR. Vorrei accennare brevemente a quelle che sono per noi le disposizioni più importanti dell'atto in esame. Riteniamo importante l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, di un tavolo tecnico per la produzione biologica, il quale avrà il compito di delineare le priorità del Piano di azione nazionale, con particolare attenzione alla ricerca. Importante è quindi l'aver previsto anche un Piano d'azione nazionale per la produzione biologica; come riteniamo importante citare le misure previste dall'articolo 6 del testo, che noi di Fratelli d'Italia sposiamo in pieno, cioè il fatto che si istituisca il marchio biologico italiano che caratterizza i nostri prodotti. Così come riteniamo importante la costituzione di distretti per la valorizzazione di zone vocate al biologico. In particolare, crediamo che questo passaggio possa aiutare le zone montane e le zone periferiche, di per sé indirizzate a pratiche di coltivazione o di allevamento naturali già per vocazione biologica (se così la possiamo definire), grazie grazie però alla scarsa industrializzazione e al basso inquinamento presenti in quelle zone. Per noi tutto quello che può valorizzare e aiutare le zone montane è positivo. Le misure che ho appena elencato sono solamente alcune nell'insieme degli interventi dell'intero provvedimento, ma sono un esempio di come il testo in esame oggi in quest'Aula vada nella giusta direzione. Il lavoro in Commissione ha profondamente mutato il testo approvato alla Camera; siamo però convinti che si poteva e si doveva fare meglio. Proprio con questo obiettivo - ad esempio - siamo intervenuti in Commissione affinché l'agricoltura biologica non fosse equiparata all'agricoltura biodinamica. Peccato per la bocciatura del nostro emendamento che chiedeva l'abolizione del comma 3 dell'articolo 1, in quanto in esso si vuole equiparare l'agricoltura biologica all'agricoltura biodinamica, indicando solo genericamente il rispetto delle disposizioni del regolamento UE in materia di agricoltura biologica, senza definire il metodo dell'agricoltura biodinamica, che - come sappiamo - è frutto solamente di autoregolazione privata e non risponde a regolamentazioni normative né europee, né nazionali. Coerentemente, abbiamo votato gli emendamenti della senatrice Cattaneo, che andavano nella stessa direzione, e ci siamo conseguentemente astenuti sugli articoli 1, 5 e 8. Abbiamo comunque dato il nostro contributo. Nella discussione in Commissione abbiamo proposto un nostro emendamento per aiutare gli agricoltori che subiscono perdite a causa della decertificazione di prodotto biologico a seguito di contaminazione durante la filiera. Come sappiamo, i prodotti agricoli italiani non possono essere venduti come biologici se presentano contaminazioni di prodotti non ammessi al sistema produttivo. Purtroppo questa contaminazione può avvenire anche durante le fasi di commercializzazione che portano il prodotto sui banchi di vendita e, quindi, dovevamo prevedere una qualche forma di ristoro. l'emendamento e abbiamo presentato un ordine del giorno condiviso che impegna il Governo ad adottare misure per compensare le eventuali perdite dei produttori. Detto tutto ciò - mi avvio alle conclusioni - credo che dobbiamo anche fare una profonda riflessione su quale potrà essere il futuro dell'agricoltura. Nei prossimi decenni la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi e il tema dell'alimentazione umana sarà al centro della discussione politica. però andare in ambiti mondiali, noi abbiamo il dovere non solo di puntare sulla qualità, ma anche di garantire un minimo di autonomia alimentare alla nostra Nazione. Già al momento abbiamo grosse difficoltà nell'essere autosufficienti in molti settori agroalimentari e nel futuro la situazione potrebbe essere ancora più critica. Non possiamo certo pensare di poter risolvere il problema puntando solo sull'incremento del biologico, senza contare poi che, sul piano sociale, rischiamo di creare anche delle discriminazioni fra cittadini che non potranno permettersi di consumare prodotti di qualità biologica a causa del loro maggior costo. Tali elementi elementi devono portarci a trovare soluzioni sempre più all'avanguardia per l'agricoltura e a coniugare produzione, modernità e qualità.

perché riteniamo opportuno dare - sì - una regolamentazione al settore tramite questo provvedimento, ma, nonostante l'enfatizzazione data al biologico, riteniamo che questa non possa essere l'unica via per la nostra agricoltura. *(Applausi)*.

recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. La mia ormai nota passione per il mondo agricolo ha condizionato e piacevolmente rivoluzionato una parte della mia vita. Quello in esame è un provvedimento importante che - lo dico subito - conferma già nella finalità la piena aderenza al sistema di regole che sono alla base del modello di produzione biologica nazionale. Non vi è alcun equivoco. L'impianto è concreto e si attribuisce all'agricoltura biologica lo *status* di agricoltura non privilegiata, ma complementare a quella che, non più definibile convenzionale, è declinata ormai come agricoltura integrata. La norma, piuttosto, entra pienamente nel solco dell'indicazione europea che vede nell'agricoltura biologica uno dei pilastri della nuova PAC, che il 25 marzo scorso la Commissione europea ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica, con l'obiettivo di aumentare produzione e consumo raggiungere il 25 per cento dei terreni agricoli coltivati con metodo bio entro il 2030, nonché aumentare significativamente l'acquacoltura biologica. In sostanza, la norma di cui oggi discutiamo contribuisce a migliorare un metodo di coltivazione - quello biologico - con mezzi che mirano a mettere in piedi un'offerta diversa. Non spetta a me, né a noi giudicare se sarà migliore o peggiore, ma è un'offerta alternativa a quella classica derivante dalla produzione agricola con protocolli integrati. E si vuole fare ciò attraverso la realizzazione di un marchio italiano di produzione biologica, la costituzione di distretti e organizzazioni di produttori e la formazione continua che guardi a veri e propri corsi di laurea; insomma, un'alternativa che tenderà a crescere e a professionalizzare nuove figure occupazionali. Non ho difficoltà ad ammettere, però, che forse la criticità del disegno di legge, soprattutto per chi lo vuole leggere solo in una direzione, è nell'iniziale enunciazione del principio di equiparazione di metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari con il metodo dell'agricoltura biologica, definendo espressamente tra questi quello dell'agricoltura biodinamica. Questo principio, tuttavia, non può estrinsecarsi nel concreto in modalità equivoche, poiché il regime della produzione biologica in Italia è rigidamente ancorato a regolamenti che ne disciplinano tutti gli aspetti, da quello delle sementi, ai metodi di produzione, fino all'etichettatura. A conferma di ciò, nel disegno di legge non si riportano mai - né potrebbe essere altrimenti - elementi specifici di applicazione concreta a tali metodi, tranne che un generico richiamo all'articolo 8 su sementi di varietà adatte anche all'agricoltura biodinamica. Gli stessi obiettivi del Piano d'azione nazionale, di cui all'articolo 7 del disegno di legge, lasciano poco spazio a elementi diversi da quelli su cui si fonda la realtà dell'agricoltura biologica in Italia. Anzi, lo specifico obiettivo di incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, specificato nell'articolo 11, conferma la direzione della norma verso un approccio inequivocabilmente scientifico. Il nuovo regolamento UE n. 848 del 2018 entrerà in applicazione tra pochi mesi e occorre da subito accelerare sulla riforma dei relativi provvedimenti nazionali o applicativi, dalla non conformità ai sistemi di controllo, all'adeguamento di acquacoltura, vino e sementi, ai sistemi di notifica, alla banca dati vigilanza, alle registrazioni obbligatorie per il sistema di controllo della produzione biologica. Tali norme applicative, con cui la nuova legge deve essere in sintonia, rafforzeranno ancora di più l'attuale impianto dell'agricoltura basato su metodi validati scientificamente, vigilati e rigidamente controllati, a garanzia del consumatore nazionale, che sta dimostrando - lo si voglia o no - una crescente fiducia verso il prodotto bio a marchio UE e che domani incrocerà il marchio nazionale a migliore presidio di un'identità produttiva, quella italiana, che tutti ci invidiano. Sarebbe un errore assistere o, peggio ancora, partecipare alla disputa biologico *versus* integrato. Io non ho le competenze per valutare le oltre 140 pubblicazioni sulla biodinamica sottoposte a referaggio su riviste scientifiche a *impact factor*, ma ho certamente il diritto-dovere da parlamentare di misurarmi con le differenti posizioni ideologiche sul modello agricolo e sugli indirizzi di sviluppo del Paese. L'approccio, però, non deve mai mettere in contrapposizione i modelli di produzione, né porre in competizione i disciplinari fitosanitari. Viceversa, nel rispetto anche del rischio di impresa che resta in capo all'imprenditore, si consente libertà di scelta al produttore, che autonomamente decide cosa e come produrre, ma anche al consumatore di scegliere. Ormai sappiamo bene - mi ripeto - che vi è sempre una maggiore attenzione nella scelta degli acquisti alimentari. Una volta si guardava velocemente solo la data di scadenza; oggi, invece, il consumatore è molto più attento: cerca i valori nutrizionali, l'origine e ogni elemento che inquadra una più sana e consapevole scelta alimentare, che è la sua. avviene nel solco di una sempre più ricercata sostenibilità ambientale, tenendo bene a mente i rischi di erosione dei suoli, l'impoverimento degli stessi per la perdita costante di sostanza organica e il rischio idrogeologico. Presidente, ho letto anch'io i recenti articoli di stampa e ho ascoltato con attenzione - come sempre faccio - l'intervento della senatrice Cattaneo, che rispetto. Proprio per questo voglio dare qui una risposta secca. Nel nostro caso l'esoterismo non c'entra nulla

Perdonatemi il parallelo che vado a fare per dire che sono tanto dalla parte della scienza che abbiamo tutti sostenuto e poi gioito per la rapidità con cui siamo arrivati al vaccino per il Covid, e con lo stesso impegno io personalmente continuo a sostenere la scienza in ogni campo, anche quando le soluzioni - ahimè - non sono così rapide e tempestive come tutti immagineremmo. Penso alla mia terra, il Salento, la Puglia, dove piangiamo ancora milioni e milioni di alberi di olivo morti a causa di un batterio da quarantena. Qui, purtroppo, la scienza non è ancora arrivata a una soluzione, ma, ciononostante, non abbiamo mai smesso di avere fiducia nella ricerca e nei ricercatori, nella scienza e nelle istituzioni, e mai abbiamo creduto ai santoni come Partito Democratico. La nostra forza sarà quella di riuscire a restare insieme per affrontare le sfide che abbiamo davanti, tenendo bene a mente i valori e gli obiettivi dell'Unione europea: solidarietà e responsabilità, promozione del benessere dei cittadini, sviluppo sostenibile e protezione dell'ambiente. È per queste motivazioni che annuncio convinto il voto del mio Gruppo Partito Democratico al provvedimento.

un ottimo lavoro su un provvedimento molto importante per il nostro Paese e per l'agricoltura italiana.

la transizione ecologica, che è diventata un punto di riferimento per la ripresa del Paese. Stiamo capendo una volta per tutte - lo spero - che ci troviamo di fronte alla necessità assoluta,

nella trasformazione i settori produttivi. In questo, l'agricoltura è un campo cruciale. L'agricoltura può dare benefici enormi sulla strada della lotta ai cambiamenti climatici, climatici, della transizione verde, oppure può dare risultati negativi se non si fa una grande operazione di accompagnamento e trasformazione. Sapete meglio di me che

un intervento complessivo che rendesse questo settore in grado di progredire ancor di più progredire ancor di più e di riuscire a essere una punta di diamante di tutta la produzione agricola. La

non sono affatto poche, è l'unica possibilità di poter avere un'agricoltura produttiva e quindi di sviluppo. Questo non lo dobbiamo dimenticare, con tutto quello che comporta, come la valorizzazione dell'identità

il *green new deal* e con gli obiettivi che ci siamo dati per l'agenda 2030 anche nei confronti dei cambiamenti climatici;

gli articoli che adesso citerò, si fa un'operazione importante ad esempio con riguardo alla questione della delega per la razionalizzazione del sistema dei controlli, del fondo, del piano strategico.

in cui questo possa svilupparsi sempre più e diventare maggiormente competitivo all'interno del mercato globale. Che cos'è il biologico? È *in primis* un metodo di produzione secondo un modello di sviluppo rurale e tutela ambientale e della salute. salute. Il metodo biologico, infatti, è sempre più centrale anche alla luce della nuova politica agricola comune, che pone come punto nevralgico il rispetto dell'ambiente e della sua sostenibilità. È stato ricordato dai colleghi che nel 2019 l'Italia si è confermata primo Paese europeo per numero di aziende agricole impegnate nel biologico, con oltre 80.000 operatori coinvolti,

La lungimiranza dei nostri agricoltori è stata premiata da consumi da *record*, con introiti pari a tre miliardi e questo senza tenere conto del comparto Horeca. Il bio costa di più ai consumatori perché - sia chiaro - costa di più al produttore agricolo, inoltre il disciplinare del bio - ricordiamolo - ha dei paletti molto stringenti entro i quali si dovranno muovere tutte le altre metodologie e produzioni, ad esempio quella della biodinamica. È necessario, però, uno sforzo maggiore, bisogna infatti anche segnalare l'incremento delle importazioni di prodotti biologici da Paesi extracomunitari, pari al più 13 quindi cercare di ridurre la nostra dipendenza e sostenere le produzioni di materia prima italiana certificata, garantendo al consumatore la qualità del prodotto e puntando così al raggiungimento di un obiettivo fondamentale della strategia *farm to fork*: il 25 per cento di superficie coltivata con metodo biologico. biologico. La questione delle materie prime oggi in particolare è il punto nodale del discorso, incidendo su ogni comparto economico-produttivo e di consumo. Assistiamo ad un incremento smisurato del costo delle materie prime, del trasporto, dei *container*, che finisce per incidere sull'aumento dei costi generali, creando serie difficoltà. Bisogna quindi lavorare per ridurre l'impatto di ciò sul sistema. Per farlo bisogna stanziare, ad esempio, le risorse necessarie anche ai nostri agricoltori, tramite il fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all'articolo 9 del disegno di legge che stiamo discutendo. Riguardo al sostegno pubblico e al comparto agricolo ciò risulta oggi più che mai vitale, visto il periodo di estrema criticità che lo stesso vive. Già prima del Covid, che ha visto la riduzione della manodopera, mettendo a rischio i raccolti, il comparto ha dovuto fronteggiare una serie di eventi: calamità naturali, diffusione di patogeni batterici, frutto anche dei cambiamenti climatici, come la xylella fastidiosa, tanto per citarne uno, che hanno prodotto danni ingenti. Tutto ciò ha costretto gli operatori, che non hanno mai interrotto la loro attività, anche a contrarre nuovi prestiti per poter garantire il prosieguo delle produzioni. Chiediamo quindi un ulteriore sforzo al Governo, oltre a quelli già effettuati - e lo faccio per il tramite del nostro sottosegretario Battistoni, che ringrazio per l'impegno e la sensibilità nei confronti del comparto dimostrati costantemente - al fine di garantire ad esempio un aiuto concreto agli imprenditori per l'accesso al credito, ad esempio rifinanziando la cambiale agraria che si è confermato un valido strumento di liquidità per le imprese del settore, soprattutto a fronte del periodo di emergenza vissuta. Suggerisco anche lo snellimento delle procedure che per via della loro complessità scoraggiano molti, molti, come un aiuto per l'accesso alle garanzie necessarie per ottenere i finanziamenti. All'interno del disegno di legge n. 988 troviamo dei riferimenti e dei rimandi che sono la sintesi perfetta di ciò che serve al comparto agricolo in generale: rafforzamento filiera, marchio biologico unico, favorire i contratti di rete, distretti biologici, monitoraggio del settore, tracciabilità. Credo sia abbastanza chiara l'importanza di ciascuna delle suddette argomentazioni.

ma bensì perché il provvedimento si presentava incompleto. Mancava una parte fondamentale e imprescindibile per Forza Italia, il tema dei controlli, che non veniva in alcun modo affrontato e, così facendo, si sarebbe fatto un danno proprio al biologico. danno proprio al biologico. Permettetemi un ringraziamento al relatore, senatore Taricco, e a tutti i colleghi della 9a Commissione per il lavoro svolto in assoluta armonia e rispetto si è svolto un ruolo importante con l'introduzione dell'articolo 19, che delega al Governo la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli. In conclusione, investire nel biologico è un approccio *win-win*, vincono le attività agricole e le attività economiche, ma vinciamo anche tutti noi, vedendo l'adozione di migliori prassi, meno impattanti da un punto di vista ambientale, per una maggiore salvaguardia delle risorse naturali. Da parte nostra però impegniamoci a tutelare il comparto, non dimenticando che l'agricoltore è anche il custode delle terre, le quali producono prodotti sani e di qualità, che tutto il mondo ci invidia. Facciamolo controllando l'operato delle aziende per tutelare chi rispetta le regole, finanziandone le attività. Alla luce dell'introduzione della normativa sui controlli, nonché del miglioramento del testo, annuncio il voto favorevole di Forza Italia.

grazie a tutti che ho seguito solo sul finale in quanto da poco membro. Un lavoro svolto in un clima costruttivo, dove ciascuno ha cercato di dare il meglio di sé per sostenere la nostra agricoltura. Tornando Tornando al provvedimento, all'articolo 1 viene definita la produzione biologica quale sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente, azione per il clima e salvaguardia delle risorse naturali. Un esempio concreto, che può far meglio capire, lo posso portare dalla mia Verona, riportando un articolo apparso sul quotidiano «la Repubblica»: Il colore simbolo è quello del rosso Amarone, ma nei 19 Comuni della Doc Valpolicella si fa sempre più largo il verde, quello della sostenibilità. È quanto emerge - alla vigilia di Anteprima Amarone - dalle rilevazioni Avepa che registra una repentina rivoluzione verde nelle aree enologiche simbolo del veronese. In pochi anni (dal 2012 a fine 2019) il biologico in vigna è infatti cresciuto del 152 per cento in termini di superficie, con un'impennata solo nell'ultimo anno di circa il 14 per cento a fronte di una media nazionale ferma nel 2019 a più uno per cento. Una tendenza bio cominciata forse un po' tardi, ma che ora non accenna a rallentare, se si considera che anche gli ettari in conversione sono cresciuti nell'ultimo anno del 10,5 a trainare i vigneti *green* Valpolicella è soprattutto il progetto RRR (riduci, risparmia, rispetta), la certificazione voluta per le aziende del consorzio a tutela dell'ambiente, prevede l'adozione di tecniche innovative in vigneto, ma anche la sostenibilità sociale e la tutela del paesaggio. Ricordo che è la prima certificazione di questo tipo in Italia. Anche qui la crescita è in doppia cifra: più 31 per cento gli ettari RRR dall'inizio della certificazione, dal 2017 a oggi. Complessivamente, in un'area di poco meno di 8.300 ettari DOP, poco meno di un quarto sono *green* o lo stanno per diventare ufficialmente dopo il periodo in conversione. Possiamo dedurre, con questo esempio, come poter tradurre gli articoli del provvedimento che stiamo discutendo. ambientale e quella per il clima vengono completamente assolte. Per quel che riguarda la salvaguardia delle risorse naturali, un importante lavoro di territorio, anche col consorzio di tutela sopracitato, si svolge in collaborazione con l'ausilio del consorzio di bonifica veronese, ente nel quale sono onorato di essere stato il rappresentante dei sindaci. Ente virtuoso, a stretto contatto con tutta la filiera agricola, al fine di preservare un bene prezioso, una risorsa naturale: l'acqua. Sia chiaro però che alimentarsi e nutrirsi con prodotti biologici è una scelta. Lo è pure produrre biologico: è una scelta

Non diventi però l'agricoltura biologica l'antitesi dell'agricoltura con metodi convenzionali. Sono due realtà che possono e devono coesistere. Ricordo che l'agricoltura convenzionale, vista la carenza di alcuni prodotti, come il grano, che talvolta dobbiamo importare, garantisce una produttività necessaria al nostro Paese.

dove continua a crescere la domanda di vini sostenibili bio». Le parole biologico, agricoltura biologica e ambiente non diventino una religione; devono essere parole legate a un contesto culturale. Una cultura che in alcuni territori del nostro Paese, anche del mio Veneto, fa raggiungere elevatissime percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti; cultura che porta sempre più a un maggior rispetto per l'ambiente. Tornando al testo del provvedimento, l'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana, contraddistinti dall'indicazione «biologico italiano»: una tutela per gli agricoltori e i produttori e una garanzia per i consumatori, visto che certificherà prodotti biologici realizzati con materie prime 100 per Tutela e difesa, nonché promozione della dieta mediterranea, del *made in italy*, in questo caso anche del marchio biologico italiano: sono questioni importantissime per il nostro Paese che ci devono accomunare, consapevoli che i nostri prodotti sono eccellenze che tutto il mondo ci invidia; coltivate, lavorate e conservate in contesti territoriali, da Nord a Sud, caratterizzati da una miriade di situazioni di microclima diversi. E non vi è prodotto che risulti uguale, spostandosi nei nostri meravigliosi territori; sapori, profumi e gusti invidiati in tutto il mondo. Da qui si deduce il motivo per il quale vi sono proposte, pratiche o leggi calate dal contesto europeo atte a depotenziare un'agricoltura e una produzione agroalimentare italiana, pietre miliari della nostra economia. Mi è piaciuta molto la reazione e la compattezza di fronte alla promozione del vino annacquato, che qualcuno vuole far passare come messaggio. Allungare il vino con l'acqua è un danno economico incalcolabile per la nostra economia agricola. È un affronto alla qualità dei nostri vini: così, all'unanimità, i componenti della Commissione agricoltura del Senato. Queste levate di scudi rendono onore alla politica italiana. Mi piacerebbe fosse sempre così ogni volta che c'è un tentativo di sabotare o scimmiottare la nostra dieta mediterranea e il *made in Italy*. È significativo che oggi ci troviamo a votare il provvedimento sull'agricoltura biologica, per coincidenza in occasione della Giornata mondiale delle api, giornata istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul ruolo fondamentale di questi insetti per l'equilibrio degli ecosistemi, la tutela dei territori e la sicurezza alimentare. Importante è la mozione presentata dal Gruppo della Lega, che impegna il Governo ad adottare interventi per la salvaguardia dell'apicoltura italiana. Quindi, sotto l'auspicio della Giornata mondiale delle api, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà favorevolmente al provvedimento relativo all'agricoltura biologica.

testo unificato approvato alla Camera nel dicembre 2018. L'Italia occupa posti di rilievo, in Europa e nel mondo, per superficie coltivata a biologico e siamo i primi per numero di operatori coinvolti nel settore. Numeri che si traducono in un vantaggio rispetto al raggiungimento del 25 per cento di superficie agricola prevista dalla strategia europea, che ora è di circa l'8,5 Visto l'incremento di superficie dedicata al biologico, l'ampia e crescente diffusione dei relativi prodotti, insieme alla necessità di adeguarsi ai regolamenti europei del 2007 e del 2018, questo disegno di legge rende necessari, per un efficace sistema di controlli e per una migliore identificazione del settore, interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. Ormai è universalmente richiesto il massimo rispetto dell'ambiente e la produzione biologica è attenta proprio a questo, per la salvaguardia del clima, della biodiversità, delle risorse naturali e di servizi ecosistemici in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Voglio chiarire, viste le polemiche giunte da vari fronti, che sono equiparati al metodo dell'agricoltura biologica solo i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica. Da qui anche la biodinamica e i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal MIPAAF con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni che ordinano Sono i consumatori a decidere sui loro acquisti, noi condanniamo soltanto cosa è dannoso e indichiamo corrette pratiche. Certamente i vegani non accetterebbero questa pratica, il biodinamico, visto che si usano parti animali. Ma questa è un'altra storia. Lavorare la terra con il metodo biologico significa utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che rispettano i cicli di vita naturali. Dopo anni di utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, ci troviamo con pochissima sostanza organica nei suoli e con una preoccupante presenza di residui di fitofarmaci nelle acque. Indispensabili, quindi, queste norme rigorose di produzione che contribuiscono innanzitutto al rispetto dell'ambiente. Da qui l'attenzione alla qualità dei prodotti e alla sicurezza alimentare, nonché al benessere degli animali. Sono previste e considerate anche pratiche virtuose, che consentano la riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dalla direttiva europea n.

tavolo è propedeutico alla stesura di un piano triennale, che ha l'obiettivo di espandere la produzione biologica, convertire piccole aziende, magari in zone svantaggiate e montane, offrire assistenza e formazione professionale, incentivare la ricerca. Il tutto con risorse attinte da un fondo già destinato. Molto importante è il riconoscimento dei distretti biologici, che vanno oltre la coltivazione genuina e l'idea di sostenibilità nel suo complesso e indirizzano tutte le attività umane verso un quadro inteso a valorizzare la bellezza del paesaggio in tutti i suoi aspetti e la conservazione dei siti naturali protetti. Centrale è l'introduzione del marchio biologico italiano, che, sulla scia dell'eccellenza che caratterizza i nostri prodotti, aggiunge valore anche in termini di economia, per un mercato contemporaneo sempre più esigente e attento. Il consumatore vuol mangiare bene e in modo etico. È un valore anche l'italianità sottolineata dal marchio, per una maggiore trasparenza sull'origine. Tutto il mondo invidia la nostra cucina e le materie prime che crescono nei nostri campi, maggiormente se contraddistinte da marchi di garanzia e di qualità a tutela del consumatore. Un marchio per un messaggio chiaro, che genera valore ed economia, che parla di rispetto della natura e della salute, di semplicità, di ritorno alla genuinità e alle tradizioni, di attenzione agli ingredienti e a ogni fase della lavorazione. In questo percorso la redditività di chi produce e chi trasforma deve essere garantita. In questo senso va la regolamentazione degli accordi di filiera e delle organizzazioni dei produttori biologici e delle sementi. di queste ultime, gli agricoltori possono produrre varietà di sementi biologiche e hanno diritto alla vendita in ambito locale e di procedere al libero scambio. Dal lungo lavoro condotto in Senato con i colleghi della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare si è giunti alla definizione dell'articolo 19, in cui si delega al Governo la revisione della normativa sui controlli per la produzione biologica, in ordine a una maggiore trasparenza delle procedure. Tra queste abbiamo inserito l'obbligo di informazione circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali. Abbiamo poi introdotto la garanzia di terzietà dei controlli, una migliore tutela dei consumatori e la revisione del sistema sanzionatorio. In conclusione, dato che, nei fatti, la coltivazione con metodo biologico riduce la produttività fino al 25 per cento rispetto alle coltivazioni convenzionali e che, d'altro canto, è stato rilevato che il 30 per cento del cibo che produciamo viene sprecato, la sostenibilità, sia ambientale che economica, del biologico, considerando il grande contributo che garantisce alla fertilità e alla biodiversità dei suoli. Fortunatamente le popolazioni stanno apprezzando sempre più il prodotto bio, tanto che negli ultimi dieci anni il consumo è più che raddoppiato. A fronte di tutto questo, pensare di continuare a consumare suolo, che sia agricolo o naturale, per cementificazioni varie, oppure di utilizzare terreni vocati all'agricoltura per sovrastarli di pannelli fotovoltaici o, ancora, di dedicare campi a coltivazioni destinate a biomassa per impianti di produzione elettrica è pura follia. Se c'è davvero una nuova consapevolezza sull'importanza del suolo agricolo e del suolo naturale, oltre che di un ambiente vivo e nel suo complesso non inquinato, è ora di dimostrarlo con politiche indirizzate a questi scopi. L'agricoltura biologica è una delle possibilità concrete che noi abbiamo. Per questo e per le ragioni che ho detto in premessa, esprimo convintamente il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Il fatto che in Commissione non ci siano stati voti contrari è segno della collaborazione che c'è stata. Voglio ringraziare il sottosegretario Battistoni e il suo predecessore L'Abbate, con con cui abbiamo collaborato molto bene. Voglio altresì ringraziare il mio predecessore, il senatore Mollame, che ha fatto gran parte del lavoro in Commissione. Grazie di cuore a tutti. Penso che il risultato sia qualcosa di buono per l'agricoltura del nostro Paese.

disegno di legge sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche; seguito dell'esame delle relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concernenti l'articolo 68 della Costituzione, non concluse nella giornata di ieri; infine, ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri. La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi nella stessa giornata di martedì 25 maggio, alle ore 14,30.

della Conferenza dei Capigruppo sono stati molto intensi, perché molte erano le questioni da trattare. Ovviamente, riferirò alla Presidente questa sua richiesta di avere un esito certo.

il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della cultura. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Signor Presidente, signor Ministro, in questo momento si parla molto di rispetto degli animali, tanto che è in discussione in 1a Commissione l'inserimento della tutela animale tra i principi fondamentali della Costituzione. È un fatto di grande importanza se si pensa che gli animali sono ancora oggi per il nostro ordinamento giuridico dei beni mobili e che l'oggetto della tutela penale non è l'animale in quanto tale, ma solo il sentimento che ha l'uomo nei suoi confronti. È di altrettanto grande importanza l'iniziativa di Paesi come Francia e Germania per mettere fine a due pratiche inaccettabili dal punto di vista della protezione animale. riferisco alla triturazione dei pulcini maschi e alla castrazione senza narcosi dei suinetti. I due Paesi hanno preso un impegno comune per sviluppare nel biennio 2020-2021 un quadro di interventi per proibire tali pratiche e individuare strade alternative, coerentemente con quanto sancito dal Regolamento europeo sull'abbattimento degli animali previo stordimento. In particolare, per i pulcini si sta lavorando alla condivisione di conoscenze scientifiche per la determinazione preventiva del sesso già in uovo. Per i suini si ragiona sull'obbligo di anestesia durante la castrazione, seguita dall'uso di analgesici per ridurre il dolore o, in alternativa, sull'immunocastrazione tramite vaccino. I Ministri dell'agricoltura dei due Paesi hanno invitato, inoltre, la Commissione europea a sostenere tale approccio, nonché gli Stati a prendere parte all'iniziativa associandosi al partenariato franco-tedesco. Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile associarsi all'iniziativa intrapresa dalla Francia e dalla Germania o quali siano, in alternativa, le misure che intende promuovere per mettere fine a queste cruenti pratiche ancora ampiamente diffuse negli allevamenti italiani.

non debbano corrispondere soltanto parole vuote, ma vi debba essere un concreto obiettivo primario di ogni singolo Paese. Ben vengano, pertanto, tutte le iniziative, anche congiunte, con gli altri Ministeri e Ministri degli altri Paesi europei per addivenire a pratiche che tutelino veramente in profondità il benessere animale nel reparto zootecnico. Nel nostro Paese c'è una preminente competenza del Ministero della salute. Risponderò, per quanto di mia competenza, dicendo che il benessere animale rappresenta il presupposto fondamentale per la produzione zootecnica sempre più sostenibile a cui concorrono una serie di fattori da presidiare contemporaneamente attraverso un approccio integrato come lo stato sanitario degli animali, gli spazi vitali a disposizione, la biosicurezza, il miglioramento genetico, le emissioni nell'ambiente e una corretta gestione dei farmaci veterinari. Il tema del benessere animale è talmente importante che entrerà a pieno titolo nella programmazione della Politica agricola comune, la nuova PAC *post* 2020. Infatti, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, permangono ancora numerosi elementi di criticità da affrontare con decisione, sia attraverso sanzioni appropriate - a fronte di comportamenti non in linea con i più elementari principi del benessere definiti a livello internazionale - sia attraverso politiche incentivanti dei processi produttivi più rispettosi dell'etologia degli animali e di interesse zootecnico. Per migliorare in modo concreto e duraturo le condizioni di benessere degli animali è necessario definire *standard* minimi significativamente superiori ai requisiti minimi stabiliti dalla legge, basati su criteri oggettivi e misurabili, in modo da indirizzare il comportamento dei vari operatori che avranno la possibilità di ottenere produzioni in grado di distinguersi sul mercato. È proprio sull'integrazione degli aspetti sanitari e zootecnici che occorre intervenire per valutare, quindi migliorare la sostenibilità delle produzioni zootecniche in linea anche con gli obiettivi della strategia *farm to fork*. Quanto ai casi specifici sollevati dagli onorevoli interroganti, si precisa che il Ministero sostiene ogni metodologia innovativa volta a permettere il sessaggio delle uova da cova in modo da destinare al ciclo riproduttivo solo i soggetti femmine precocemente individuati. La metodologia oggi disponibile messa a punto da una *joint venture* tra l'Università di Lipsia e una catena di supermercati tedesca, oltre ad essere molto costosa, ha, però, bisogno di essere ulteriormente testata prima di essere applicata su vasta scala. Per quanto concerne, invece, la pratica della castrazione dei suinetti, sono in fase di definizione disciplinari produttivi contenenti impegni concreti, come comunicatoci dal Ministero della salute, al fine di superare definitivamente il problema sollevato dagli onorevoli interroganti. Il sistema unitario di certificazione del benessere animale a cui stiamo lavorando accelererà la fase di transizione del sistema produttivo. In ogni caso, assicuro che sarà seguita con la massima attenzione l'evoluzione della sperimentazione, anche al fine di definire specifici strumenti di supporto da mettere a disposizione del sistema produttivo. Stiamo inoltre valutando di inserire - nei vari incentivi per il settore zootecnico erogati dal Ministero - delle premialità per le imprese che operano nel rispetto del benessere animale. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Unterberger,

Spero che il Governo possa appoggiare questo mio disegno di legge.

Gentile Ministro, oggi, grazie al *question time*, ho l'occasione di rappresentarle una questione molto delicata che riguarda, sì, l'agricoltura, ma anche il rilancio del dialogo per la definizione di una prospettiva più ampia del sistema Paese. Con una sua nota del 23 marzo 2021 indirizzata alla Conferenza Stato-Regioni, al fine di acquisire l'intesa ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, è stata avanzata la proposta di ripartizione dei fondi assegnati all'Italia nel settore dello sviluppo rurale: il cosiddetto FEASR per gli anni 2021 e 2022, periodo transitorio determinato dallo slittamento della programmazione 2021-2027, che sarà avviata a partire dal 2023 a causa del Covid. In particolare, si propone di cambiare i criteri di ripartizione del FEASR per gli anni 2021 e 2022, passando quindi dai criteri storici a criteri oggettivi in quanto in grado di allocare le risorse in maniera equa, paragonati all'applicazione delle risorse assegnate per il *de minimis*. Signor Ministro, mi permetta di dirle che la proposta di rimodulare con nuovi criteri i fondi europei per lo sviluppo rurale, già destinati alle Regioni del Mezzogiorno, è inaccettabile sia dal punto di vista sociale che economico. Se venisse confermata questa rimodulazione, saremmo davanti ad una penalizzazione mortificante per Regioni già svantaggiate che, paradossalmente, sarebbero private proprio dei fondi destinati a garantire il riequilibrio strutturale, a tutto vantaggio di zone già di per sé meglio attrezzate. L'agricoltura è un settore strategico per le Regioni meridionali e vanno sostenute le imprese e i fondi dei Signor Ministro, le chiedo se intende trovare una soluzione condivisa con le Regioni del Sud sui criteri di ripartizione dei fondi europei per l'agricoltura e se inoltre non ritenga opportuno insediare un tavolo tecnico a cui demandare la definizione, entro sessanta giorni, dei parametri da applicare dal 2023, cercando di applicare criteri coerenti allo spirito e alle finalità del PSR.

esattamente nella misura in cui sono stati esposti anche nella domanda dell'interrogante. Alla proposta che abbiamo fatto a marzo ha fatto seguito poi una proposta del 21 aprile, che recava un'ulteriore rimodulazione rispetto al rapporto tra criteri oggettivi, nuovi criteri e criteri storici. Posto questo, vorrei fare alcune considerazioni sia di metodo che di merito, partendo dal 16 gennaio 2014 quando, dopo una discussione accesa (parliamo di sette anni fa), di sette anni fa), le Regioni avevano concordemente definito il settennato 2014-2020 come l'ultimo di applicazione dei criteri cosiddetti storici, per poi arrivare nel 2021 alla definizione di nuovi criteri. Il dibattito è nato alla fine dell'anno scorso e non ha portato a una condivisione da parte delle Regioni. C'è un blocco di sei Regioni del Centro-Sud (perché l'Umbria non è certamente del Sud, non c'è una divisione Nord-Sud in questo senso)

in un biennio, su un importo complessivo del fondo di 3,5 miliardi. Credo quindi che occorra anche dare il giusto peso alle cifre. Ovviamente è evidente che il FEASR è uno strumento molto importante per l'agricoltura italiana, in particolare per le aree in via di sviluppo agricolo, che hanno bisogno di sviluppo agricolo, ma non è l'unico strumento. Dobbiamo lavorare sulle percentuali di cofinanziamento, dobbiamo lavorare fortemente sul primo pilastro con il percorso di convergenza interna; dobbiamo dare anche molti altri strumenti a quelle Regioni per sviluppare l'agricoltura nelle aree rurali e credo che complessivamente gli strumenti che mettiamo a disposizione, anche e soprattutto delle Regioni del Sud,

applicando questi nuovi criteri addirittura alla Sicilia sarebbero stati decurtati circa 100 milioni di euro, mentre alla Campania, alla Puglia, alla Basilicata, alla Calabria e all'Umbria altri 300-400 milioni di euro. Mi rendo conto che sono cifre davvero preoccupanti. Tra l'altro, signor Ministro, stiamo cercando di uscire faticosamente da una crisi che è prima di tutto sanitaria e poi economica, ma che ormai è diventata una crisi sociale a tutti gli effetti. Decurtare ancora di più le cifre a favore dell'agricoltura

penso nel testo scritto sia ampiamente documentata e circostanziata. Sta di fatto che tra la seconda metà di marzo e la prima metà di aprile di quest'anno l'intero territorio nazionale

del 29 marzo 2004, n. 102. Tutti gli anni, quindi, come parlamentari, cerchiamo di recuperare le risorse per far fronte a questi danni e dare ristoro agli agricoltori che li hanno subiti. Credo che questo non sia il modo giusto per affrontare il problema, dobbiamo trovare una soluzione strutturale. Siamo qui non solo per recuperare le risorse nei casi di emergenza, ma per valutare quali sono le misure che dobbiamo mettere in campo affinché a fronte di eventi che possono capitare tutti gli anni, ci siano gli strumenti che pongono dei rimedi. il tema delle assicurazioni c'entri con questo tipo di problema e che debba essere preso in considerazione per trovare delle forme strutturali per affrontarle. È evidente che in agricoltura non pensiamo solamente al ristoro dei danni, ma c'è tutta una filiera che ha necessità del prodotto da lavorare, quindi la difesa attiva

un ulteriore aspetto. È indispensabile introdurre clausole di salvaguardia che limitino la riduzione della VPC e delle risorse comunitarie dei programmi operativi negli anni successivi a quelli in cui si sono verificati tali eventi: i prodotti e ha fatto programmi operativi, necessariamente messi in difficoltà dagli eventi climatici negli anni successivi, rischia di non godere delle agevolazioni alle quali aveva avuto accesso.

gli effetti dei cambiamenti climatici ci saranno ancora per un po' in agricoltura. È chiaro poi che la questione assicurativa è centrale, nel senso che è un po' un cane che si morde la coda, se vogliamo dirla così. Poche aziende si assicurano, i prodotti delle compagnie sono quindi più rischiosi e meno attrattivi, con premi più alti e fatti in campagne assicurative nei periodi sbagliati dell'anno. Il prodotto non è quindi eccezionale e le aziende continuano a non assicurarsi. In tutto questo si inserisce poi la deroga al che in qualche modo dà quella garanzia di ristoro; forse bisognerebbe trovare il modo per interrompere questo circuito vizioso. Stiamo lavorando per aumentare il prelievo dall'1 al 3 per cento per la gestione del rischio, come abbiamo proposto in sede europea a tutti gli altri Stati membri. Speriamo di ottenere un risultato proprio per aumentare la dotazione del fondo di mutualizzazione così da poter garantire la copertura delle spese assicurative in modo più proficuo per l'azienda, anche se i limiti di percentuale oggi non ci consentono di arrivare, come proposto dagli interroganti, all'80 per cento, essendo al limite massimo del 70 quanto riguarda la possibilità di incrementare lo stanziamento di risorse del Fondo di solidarietà nazionale, utilizzando anche le risorse della PAC relativa al prossimo periodo di programmazione, rammento che i nuovi fondi unionali relativi entrambi ai pilastri della PAC saranno gestiti in modo integrato attraverso un unico piano strategico nazionale e questo sarà anche un vantaggio. L'obiettivo è di perseguire un maggiore coordinamento tra i diversi tipi di interventi che concorrono alla fase di prevenzione e mitigazione dei rischi, al fine di minimizzare la probabilità del verificarsi di eventi che possano determinare la necessità di successivi interventi per ripristino ad indennizzo *ex post*. Per quanto concerne la necessità di rafforzare e promuovere i fondi mutualistici in grado di compensare finanziariamente gli agricoltori e gli allevatori per le perdite, come ad esempio inquinamento, contaminazione, malattie e qualità dell'ambiente connessa ad un determinato evento di portata geografica limitata, evidenzio che nel corrente periodo di programmazione è stata data priorità ai soli fondi per rischi climatici e sanitari, escludendo nella fase iniziale di attivazione i fondi per le emergenze ambientali. Al riguardo sono già stati riconosciuti ufficialmente quattro fondi di mutualità contro le fitopatie, le infestazioni parassitarie e, al contempo, per agevolare la fase di riconoscimento, sono state emanate apposite linee guida dedicate a possibili proponenti e fondi di mutualità. Entro l'anno è prevista l'adozione del preavviso pubblico per la corresponsione del sostegno nell'ambito della sottomisura 17.2 del Programma di sviluppo rurale nazionale. Pertanto, anche nel nuovo periodo di programmazione, è stato confermato il sostegno ai fondi di mutualizzazione. Inoltre si fa anche un lavoro di informazione presso le aziende agricole, proprio per stimolare le assicurazioni. Concludo dicendo che nel disegno di legge che abbiamo approvato pochi minuti fa è previsto il finanziamento in base al decreto legislativo n. 102 per 105 milioni di euro, un importo oggettivamente importante, uno dei più grandi importi che siano mai stati

nella sua compiutezza, proprio alla luce della considerazione da cui è partito il Ministro; non possiamo immaginare un'agricoltura che ogni due o tre anni perde di fatto un raccolto; soprattutto nelle realtà dove il tasso di assicurati sul totale degli agricoltori è molto basso, ciò rischia di essere devastante per l'agricoltura. Tra i tanti punti che abbiamo posto nell'interrogazione, mi permetto di riprenderne uno: credo sia arrivato il momento di aprire una seria riflessione

come succede adesso anche due o tre volte in un decennio, perdono completamente un raccolto. Non è sostenibile in questa stagione. Quindi, piuttosto che mettere ogni due o tre anni 100 o 200 milioni sul Fondo di solidarietà nazionale,

Signor Presidente, sono passati tre anni dal crollo del ponte Morandi e, dopo il miracolo compiuto

perché non vi è nessuna vera capacità di preordinare i lavori, quando necessari per la sicurezza, secondo le priorità e con l'accordo dei Comuni. La situazione è veramente drammatica

delle aziende turistiche, dei turisti, dei genovesi e dei liguri? La Liguria è terzo mondo in fatto di viabilità in questo momento. Ripetutamente,

chiesto risposte, ma non abbiamo ancora ottenuto risposta neanche alla prima interrogazione di più di un anno fa. Chiediamo sia considerata prioritaria la situazione della viabilità in Liguria e che il Governo ci metta la testa e dia risposte, non solo a parole.

Questo Governo ha già avviato, attraverso le strutture ministeriali competenti, un monitoraggio molto attento dello stato dei ponti e dei viadotti, non solo in Liguria, ma anche in altre parti del Paese, definendo le linee di azione e programmando interventi manutentivi. In particolare, sono state impartite specifiche indicazioni ai gestori stradali e autostradali, finalizzate a innalzare gli *standard* di sicurezza delle infrastrutture e a rafforzare la qualità e la quantità dei controlli. Al contempo, al fine di rafforzare i controlli in materia di sicurezza, sono in corso nuove iniziative, anche di natura legislativa, per definire in modo compiuto le attività e le funzioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), alla cui direzione proprio oggi, dopo la decisione del Consiglio dei ministri, è stato preposto l'ingegnere Domenico De Bartolomeo. Relativamente alle ispezioni e agli interventi di riqualificazione e adeguamento in corso lungo la rete autostradale della Liguria, che certamente anche per noi è una priorità importante nella discussione con la competente Commissione, anche in vista di futuri commissariamenti, evidenzio che si tratta di attività necessarie per la cui effettuazione il Ministero intrattiene costanti interlocuzioni con il concessionario per individuare, d'intesa con la Regione e gli enti locali, le modalità più idonee a garantire la massima riduzione dei disagi per l'utenza. Proprio a seguito della situazione del viadotto Valle Ragone è stato creato un luogo di coordinamento con gli enti territoriali e le principali associazioni di categoria, nell'ambito del quale periodicamente si condividono i programmi di intervento e le misure di ottimizzazione del traffico. Con specifico riguardo proprio al viadotto citato, evidenzio che il 12 maggio scorso, a seguito di una verifica straordinaria eseguita sull'autostrada A12, il concessionario ha disposto in via prudenziale il divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia dei mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. Detta limitazione è stata eliminata in data 15 maggio, a seguito dell'effettuazione di interventi di ripristino. Quindi vorrei confermare che il Governo sta seguendo con molta attenzione questa tematica, in particolare per ciò che riguarda la Regione Liguria.

per tutta la stagione turistica, il traffico sulle autostrade, ma persino sulla via Aurelia dove ci sono piccole frane che non vengono aggiustate e si procede a senso unico alternato con alcuni semafori posticci che vengono messi all'uopo, è rimasto lo stesso. Le parole non ci convincono. Vorremmo i fatti. Vorremmo, per esempio, che il Governo dicesse che, come ristoro, per tutta l'estate non si pagherà il pedaggio per autostrade che non sono autostrade ma strade a senso unico, con entrate e uscite da un lato all'altro, sfrecciano a pochi centimetri dalle macchine, con incidenti e tamponamenti continui. Le parole lasciano il tempo che trovano. I liguri e i cittadini italiani e stranieri che vogliono raggiungere la Liguria hanno bisogno di fatti, non di parole e di coordinamento delle autostrade e delle autorità preposte con i sindaci della Liguria, cosa che non avviene. Me lo conferma il sindaco di Rapallo con cui ho parlato poco tempo fa. La ringrazio per la sua cortesia, ma sono comunque assolutamente scontento delle iniziative che il Governo non prende per ovviare all'enorme disagio della viabilità in Liguria.

È assolutamente indispensabile lo sviluppo delle infrastrutture per essere competitivi in tutti i settori economici, nell'industria, nell'agricoltura, nel turismo e in tutti i settori economici del nostro Paese. In questo, lo sviluppo dei treni ad alta velocità che oggi consentono di spostarsi con grande rapidità in molta parte del Paese, non in tutto, è stata sicuramente un'iniziativa per la quale nutriamo particolare orgoglio, essendo stata portata avanti dal Governo Berlusconi, in particolare dal secondo e dal terzo. Ora vengono Ora vengono impegnate grandi somme del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in questo settore. Tuttavia, abbiamo letto con una certa preoccupazione alcune sue dichiarazioni riguardanti il ponte sullo Stretto di Messina, che è vero che non risolve evidentemente i problemi di viabilità generali della Sicilia, ma indubbiamente, se non c'è modo di arrivare rapidamente in Sicilia, è molto difficile pensare a un miglioramento delle autostrade di quella Regione. Allo stesso tempo abbiamo letto delle dichiarazioni, da lei rilasciate alla stampa il 12 maggio, sulla linea ad alta capacità, sebbene oggi sia ancora conosciuta come linea ad alta velocità, Torino-Lione.

linee che ho elencato: Liguria-Alpi, Palermo- Catania-Messina, Napoli-Bari, Verona-Brennero, Roma-Pescara, Orte-Falconara, Taranto-Battipaglia e Salerno-Reggio Calabria.

dopo la trasmissione al Parlamento della relazione finale del gruppo di lavoro tecnico per la valutazione di soluzioni alternative, il Governo considera assolutamente fondamentale il confronto con il Parlamento, con le altre istituzioni e con la società civile, in modo da poter avere l'adozione di una decisione, che consenta di rispondere al meglio alla domanda di mobilità da e per la Sicilia, con infrastrutture e mezzi di trasporto adeguati e sostenibili sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Vorrei ricordare - - ciò non vuol dire che la discussione si chiude, tutt'altro - che nel PNRR sono comunque inseriti importanti investimenti, che riguardano l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina e l'attraversamento dinamico dello Stretto, in maniera tale da migliorare, nel frattempo, la situazione dei cittadini e, naturalmente, delle imprese. In merito alla tratta europea della TAV, l'opera è in esecuzione, in virtù di un accordo internazionale approvato dal Parlamento e, con la sottoscrizione, nell'aprile 2020, dell'*amendment* al contratto di sovvenzione europea, il finanziamento comunitario è stato integralmente conservato, con un'estensione temporale a tutto il 2022. Per la tratta nazionale sottolineo assolutamente l'importanza dell'opera, ma sappiamo anche che, visto che che RFI non ha effettuato la progettazione di una parte della tratta nazionale, serve un confronto con i territori e di questo ho parlato anche nella mia intervista, in maniera tale da poter procedere prima possibile alla progettazione della tratta nazionale. Segnalo infine che sono in via di definizione le nuove nomine di competenza del Governo italiano nel consiglio di amministrazione della TELT-Tunnel Euralpin Lyon Turin, nel comitato di controllo e nella commissione contratti. Quanto ai progetti ad alta velocità e alta capacità Liguria-Alpi, Palermo-Catania-Messina, Napoli-Bari, Verona-Brennero, Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto-Battipaglia, evidenzio che sono tutti interventi inclusi nel PNRR, la cui realizzazione avverrà secondo il cronoprogramma inserito nel piano, che, come noto, è ora all'attenzione della Commissione europea, per l'approvazione definitiva. In ogni caso, gli interventi citati dovranno essere completati entro il 2026, come previsto dal Next generation EU. realizzazioni, il cui completamento è previsto entro il 2030. Anche nel PNRR, però, ci sono interventi per alcune tratte della Salerno-Reggio Calabria, come sappiamo, e una parte della Brescia-Vicenza-Padova è già in esecuzione, come ricordato recentemente anche da Ferrovie dello Stato. Per ciò che concerne la Sardegna, che pure non è oggetto dell'interrogazione, le stiamo prestando un'attenzione particolare nel PNRR;

La ringrazio, signor Ministro, per le rassicurazioni e i tempi di cui ci ha parlato. Ha aggiunto anche il tema delle nomine per determinate società, che sono fondamentali per la realizzazione di quanto il nostro Paese necessita. Conto che tali nomine siano fatte con il criterio della competenza e della condivisione della necessità, per il nostro Paese, di completare queste opere,

l'attraversamento dello Stretto di Messina, lei ha parlato di attraversamento stabile e di attraversamento dinamico. Sarei stato più rassicurato se avesse detto la parola "ponte"; però, se la sostanza è quella, va bene. Sappia che

possibilità economiche, degli scambi e degli spostamenti nelle zone del nostro Paese che sono state toccate dall'alta velocità ferroviaria, oltre naturalmente alla necessità di provvedere anche negli altri settori delle infrastrutture.

Signor Presidente, ringrazio il Ministro per l'attenzione. Come noto, nell'aprile 2020 sono state emanate le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di sorveglianza di ponti e viadotti, costituiscono il riferimento per l'adozione, da parte di Anas e dei concessionari autostradali, delle azioni da porre in essere in ordine all'approfondimento e alla frequenza delle ispezioni, alla programmazione temporale degli interventi, nonché agli eventuali provvedimenti di limitazione del traffico. Tuttavia, sappiamo che i ritardi burocratici incidono molto sulla programmazione e sull'esecuzione degli interventi di manutenzione obbligatoria a cui devono essere sottoposti i viadotti in base ai parametri stabiliti dalle linee guida in questione. Quindi, considerato che le ispezioni da parte del personale del Ministero possono determinare la chiusura immediata di intere tratte autostradali che presentano criticità a causa di ritardi nella manutenzione - come citato poc'anzi questo meccanismo può creare vere e proprie distorsioni, anche con l'adozione improvvisa di provvedimenti di limitazione del traffico in seguito a sopralluoghi da parte del Ministero e di Aspi (com'è accaduto nel caso del viadotto di Valle Ragone, che abbiamo sentito esporre poc'anzi da un altro senatore interrogante), dobbiamo tuttavia ricordare in quest'ambito che i sindaci dell'area inerente al viadotto di Valle Ragone avevano già chiesto e segnalato più volte ad Autostrade per l'Italia la necessità di un controllo della zona relativa. Questo Questo è avvenuto anche nel febbraio 2021. È stato risposto a questi sindaci, che lavoravano in sinergia, che i controlli sono trimestrali e quindi non è stato seguito un approccio costruttivo nei confronti dei sindaci del territorio (questo è motivo di rammarico). Considerato che ormai sono passati tre anni dalla tragedia del ponte Morandi, purtroppo non esiste ancora un piano che garantisca una compatibilità tra gli interventi di messa in sicurezza delle opere e le esigenze di imprese e cittadini. Queste misure di blocco improvviso penalizzano infatti soprattutto i trasporti eccezionali, creando grandi danni economici a tutti gli operatori del settore. Tale situazione però rischia soprattutto di sfavorire tutti i cittadini e le imprese che usufruiscono del trasporto su gomma, causando code e rallentamenti dovuti allo spostamento obbligato dei mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria. Tutto ciò premesso, con quest'interrogazione sollecitiamo il Governo per sapere quali iniziative di propria competenza intenda adottare per modificare questo meccanismo di chiusura improvvisa di autostrade importanti, chiarendo anche il criterio in base al quale sono scelte le arterie oggetto di ispezione, al fine di garantire una compatibilità tra gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture e l'esercizio di tutte le attività economiche, compresa quella dei trasporti eccezionali.

Dobbiamo però renderci conto che nei prossimi anni l'Italia dovrà impegnare rilevantissime risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, in un'ottica di prevenzione dei rischi, considerati il prevedibile impatto dei cambiamenti climatici, ma soprattutto la vetustà di alcune opere. Personalmente nel 2009 guidai, all'OCSE, un gruppo di ricerca che mostrò come, intorno agli anni 2020-2030, tutti i Paesi industrializzati che avevano costruito le proprie infrastrutture nel Secondo dopoguerra avrebbero dovuto fronteggiare problemi e soprattutto spese molto rilevanti per metterle in sicurezza. Ovviamente, una delle iniziative fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del Paese, ma anche in chiave di sostenibilità, è la messa in sicurezza delle nostre infrastrutture, che devono corrispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede, proprio per questo settore, un investimento senza precedenti, a cui si sommano anche gli investimenti sui fondi nazionali. Naturalmente, nel breve termine i disagi ci sono. Venendo alla rete stradale e autostradale ligure, sono in corso diversi interventi di riqualificazione e adeguamento, incentrati particolarmente su viadotti, ponti, gallerie, barriere e protezioni acustiche.

Su specifica richiesta del Ministero, i gestori hanno avviato indagini per accrescere la conoscenza dello stato delle singole infrastrutture e per una migliore programmazione degli interventi di manutenzione, così da ridurre al massimo il disagio all'utenza. Proprio per questo, dopo l'evento che lei ha citato, è stato attivato un tavolo di coordinamento con gli enti territoriali e le principali associazioni di categoria, nell'ambito del quale si condividono i programmi di intervento e le misure di ottimizzazione del traffico. Visti l'orientamento al turismo della Liguria e la prossima stagione estiva, bisognerà contemperare le diverse esigenze In merito al meccanismo di scelta delle arterie oggetto di ispezione, gli interventi vengono effettuati sulla base dei criteri indicati nelle linee guida. Da questo punto di vista, il Ministero ne segue attentamente Con la circolare del Ministero del 9 aprile ultimo scorso è stato inoltre predisposto un piano di sorveglianza da applicare a ciascuna galleria, in modo tale da realizzare interventi programmati in anticipo. Le nuove linee guida adottate, nonché la citata circolare impongono ai gestori (ivi compresa Anas) di effettuare un'attività di vigilanza secondo modalità stringenti, che consentano di acquisire un profondo stato di conoscenza delle infrastrutture e riducano al minimo il rischio di rilevare criticità improvvise, il cui superamento potrebbe imporre l'adozione di misure straordinarie sulla circolazione. In conclusione, proprio per ciò che concerne le attività di manutenzione delle strade statali, Anas esegue procedure standardizzate di controllo su tutte le opere d'arte, con quattro ispezioni ricorrenti trimestrali e una più approfondita una volta l'anno.

Sono molto contento che prima abbia citato la nomina del nuovo presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali, perché purtroppo è rimasta per circa per quasi due anni, da quando venne lanciata dall'allora ministro Toninelli. Di sicuro, auspico che il nuovo presidente riesca a rilanciare e strutturare quest'agenzia per riuscire a ottenere dei risultati a breve tangibili e misurabili. Oggi abbiamo la Liguria come punto di riferimento, che ha sofferto in prima persona e sta soffrendo un grande disagio, però, da montanaro dell'Appennino modenese, devo dire che il problema della viabilità sentito in maniera trasversale in tutto l'Appennino e non solo. Mi auguro che si possa fare un buon lavoro insieme. Siamo sempre a disposizione - lo abbiamo dimostrato - per essere di aiuto al suo Ministero e collaborare in maniera fattiva.

la gestione del personale in seno al Ministero della cultura è, da tempo, un punto molto dolente. Tagliata la pianta organica da circa 25.000 a circa 19.000 unità, stante la combinazione di pensionamenti massivi e blocco del *turnover*, restano in servizio effettivo poco più di 12.000 dipendenti, con lacune gravissime in tutti i ruoli.

limitatamente alle procedure in atto, il concorso bandito nel 2019 per 1.052 posti di addetti alla fruizione accoglienza e vigilanza (AFAV) è fermo da quasi due anni.

(per accelerare, invece che in modalità decentrata, si potrebbe pensare di tenerlo a Roma in simultanea), né sanno se, superato quello, saranno chiamati a sostenere la prova orale come previsto nel bando. A quest'ultima si potrebbe rinunciare, in tempo di pandemia, tanto più che la conoscenza di CAD e ITC e la padronanza della lingua inglese saranno accertate nello scritto, e soprattutto in considerazione della drammatica carenza di personale del la selezione indetta, invece, il 29 dicembre 2020 per le collaborazioni a contratto con le Soprintendenze ABAP, *ex* art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 di 500 professionisti (archeologi, architetti, storici dell'arte, ingegneri, assistenti di cantiere e tecnici contabili) tocca, a parere dell'interrogante, vertici di scorrettezza senza precedenti; anomalie si rinvengono già nell'avviso di selezione, poi nelle liste provvisorie dei vincitori e degli idonei ricavate dalle 2.138 istanze pervenute, nella comunicazione che procrastina l'ostensione degli atti per i moltissimi presunti non idonei, che hanno fatto istanza, nella mancata richiesta del *curriculum*, nella ripartizione dei punteggi e altro, si chiede di sapere: a proposito del concorso per 1.052 AFAV, se il Ministro in indirizzo sia in grado di indicare una data certa per lo svolgimento della prova scritta, confermare o meno la prova orale e illustrare un cronoprogramma ragionevolmente preciso in ordine alla tempistica dell'intera procedura; a proposito della selezione dei 500 collaboratori delle Soprintendenze ABAP, se il Ministro non ravvisi l'opportunità di un'immediata sospensione e revoca di detta selezione, anche per i profili di danno erariale prevedibili in ragione dei contenziosi ai quali si apre la strada, nonché la necessità del contestuale avvio di una più rapida, coerente ed economicamente vantaggiosa procedura di internalizzazione delle figure professionali dipendenti dalla società *in house* ALES

in relazione al concorso per 1.052 AFAV, la prova scritta è stata procrastinata, come per tutti i concorsi *in itinere*, a seguito dell'emergenza sanitaria. Già nel corso del 2020 il Ministero, ferma restando l'esigenza primaria di salvaguardare la tutela della salute dei candidati, come per tutti gli altri concorsi, e del personale impegnato nelle attività di vigilanza, ha chiesto al Formez, del cui supporto si avvale la commissione interministeriale per l'attivazione del progetto di procedere al riavvio della procedura concorsuale con la calendarizzazione della prova scritta, anche avvalendosi delle modalità di svolgimento delle nuove prove previste dall'articolo 248 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per la prova scritta e modalità in videoconferenza per le prove orali. Di questo stiamo concludendo - con il competente Dipartimento della funzione pubblica - le modalità di svolgimento. Relativamente alla cosiddetta selezione dei 500, la direzione generale competente ha avviato - nel dicembre 2020 - la procedura comparativa per soli titoli e requisiti professionali per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi della norma di legge. Non si tratta - voglio specificarlo, perché ho letto qualcosa sui giornali - di un concorso pubblico, ma di una procedura da espletarsi in tempi rapidi, tenendo conto della scadenza per lo svolgimento degli incarichi, attraverso cui individuare non dipendenti nuovi, ma professionisti di supporto agli uffici e non reclutare quindi personale interno. Si è dunque deciso che la domanda di partecipazione, redatta secondo il *format* messo a disposizione del Ministero sulla piattaforma informatica, dovesse essere corredata da una sintetica presentazione personale, con l'indicazione dei titoli di studio conseguiti e delle esperienze professionali maturate, autodichiarati dal candidato, sufficienti a rappresentare in maniera efficace la formazione acquisita con corsi di alta formazione, perfezionamento scientifico e aggiornamento, nonché le esperienze professionali ritenute rilevanti e qualificanti per una competenza peculiare nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio. Sono arrivate 2.138 istanze, che sono state valutate da una commissione composta esclusivamente da dirigenti del Ministero, così come riportato nell'avviso di selezione, che ha considerato per ciascun candidato l'esperienza professionale maturata, la specifica formazione e la lettera motivazionale presentata.

a cui gli stessi sono assegnati. Voglio ulteriormente sottolineare che l'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata all'esito del controllo preventivo della Corte dei conti. Quindi, per tutti questi motivi e proprio per l'esigenza di personale che lei stessa

*(Misto)*. Signor Ministro, sa, non mi aspettavo di vederla qui oggi. Ero convinta di dover replicare alla sua ombra, al suo cenere muto, quindi averla in presenza mi permette invece di correggere un errore che ho commesso nell'ultima occasione in cui ci siamo trovati nelle stesse circostanze, quando le dissi che sarebbe stato ricordato come il peggiore Ministro dei beni culturali della storia della Repubblica. Nel frattempo, ha cancellato i beni culturali persino dalla denominazione del suo Ministero, quindi questo mi ha aiutato a riflettere e mi ha fatto capire l'errore, e cioè che l'ho sottovalutata e ho sottovalutato la sua ambizione, ben più alta: evidentemente, aspira a salire al Colle, nell'una o nell'altra veste, proprio grazie a quei demeriti che, in ogni caso, le consentiranno di essere ricordato semplicemente come il peggiore Ministro della storia della Repubblica e punto, (e questa palma credo non gliela tolga nessuno). Mi riesce veramente difficile capire come abbia potuto - anche presso i *media* - accreditarsi come un fine politico. In realtà, solo in un Paese soggiogato da un provincialismo e da una mediocrità costanti è possibile un ribaltamento dei valori tale per cui la politica, invece che essere servizio, diventa una sorta di tessitura di trame e di scambio di favori personali con portatori di interessi. Lei ha risposto sui 1.052 AFAV, dando una risposta che, a mio avviso, è un vero e proprio gioco di prestigio,

parlavo della procedura dei 500. La risposta è un affronto all'intelligenza collettiva e vorrei accennare alla lettera che alcuni di costoro - come sa, signor Ministro - hanno mandato al Presidente della Repubblica, mantenendola però riservata, per pudore, il che non significa che abbiano timore di ritorsioni, ma che si vergognano, di lei e della situazione. Parliamo di professionisti plurititolati che collaborano da anni con la burocrazia creativa del suo Ministero e che però sono stati per l'ennesima volta, presi in giro e maltrattati.

oltre all'emergenza pandemica che stiamo affrontando da un anno, sullo sfondo, sempre più incombente, ce n'è una climatica, che necessita di un vero cambio di paradigma, che ponga al centro delle decisioni politiche il benessere del pianeta e delle persone.

legati ai cambiamenti climatici, se è vero che entro il 2050 ci dobbiamo aspettare un innalzamento dei mari di 20 centimetri e se pensiamo anche a tutti i fenomeni di dissesto idrogeologico che si vanno aggravando nelle parti interne del nostro Paese. Nel Piano nazionale di ripresa e risorse; mi lasci dire che potevamo fare di più, soprattutto riguardo alle attività di manutenzione programmata, preventiva e ordinaria. Sa bene che sono numerose le critiche mosse dai professionisti del comparto rispetto agli annosi problemi del settore: non si tratta solo di un'assenza di pianificazione e di fondi per la gestione ordinaria, ma di carenza di personale, prospettata sospensione delle attività di archeologia preventiva, come denunciano alcuni professionisti in un articolo de «il Fatto Quotidiano» del 19 maggio (quindi è recentissimo), perenne esternalizzazione dei servizi e assenza di un'attività di mappatura completa. Sa bene che lo stringente cronoprogramma del Governo per mettere in campo gli appalti *green* rischia di mettere in difficoltà gli organismi che già si trovano sotto organico e sono colpiti da una riforma della loro organizzazione (quella del 2014) che ha fortemente penalizzato la loro efficienza e la loro efficacia. Non si tratta quindi di fare barricate, tuttavia, signor Ministro, le chiedo quali iniziative intenda assumere in merito al prossimo decreto-legge semplificazioni, tenuto conto del principio costituzionale della tutela del patrimonio, e quali iniziative intenda intraprendere al fine di risolvere queste annose criticità e i gravi problemi riferiti all'organizzazione e alla carenza di organico, soprattutto all'interno delle sovrintendenze.

rendono più agevole e tolgono gli intoppi per rispettare i tempi, ma in generale, perché bisogna dare risposte alle istanze del mondo produttivo e dei cittadini, senza però indebolire i principi di tutela. Su questo credo che all'interno del Governo stiamo raggiungendo un equilibrio che il Parlamento potrà Stiamo ragionando anche di misure straordinarie, come ad esempio l'ipotesi che per le opere del PNRR ci sia una soprintendenza unica nazionale che vale per le opere che attraversano le competenze territoriali di più soprintendenze, come capita per una grande infrastruttura o per quelle che superano un determinato valore, sempre nell'idea

e soprattutto è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il principio del corso-concorso per i dirigenti tecnici del Ministero, che è già stato bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività

di una transizione ecologica. Non sono soddisfatta, signor Ministro, perché non sono assolutamente convinta che la riforma delle sovrintendenze abbia portato aspetti positivi, ma non sono io a dirlo, bensì gli operatori stessi che operano ogni giorno in tutti i cantieri all'interno delle sovrintendenze. Le chiedo quindi di fare un ulteriore sforzo e di leggere con attenzione l'articolo che richiamavo de «il Fatto Quotidiano», ma anche quanto scrive oggi Andrea Carandini, presidente del FAI, in un intervento in cui le pone in modo molto chiaro, sintetico, ma incisivo, alcune questioni, tra cui anche quella della sovrintendenza

con animo sereno, pensando al bene di questo Paese e del suo patrimonio artistico e paesaggistico, una quadra tra le esigenze di un cambio di paradigma in una direzione di ecologia e di decarbonizzazione

durante l'esposizione della senatrice Corrado, perché voglio che sia lasciato agli atti che non è possibile utilizzare in quest'Aula in quest'Aula le espressioni che la senatrice ha usato, che vanno assolutamente al di fuori del contenuto dell'interrogazione formulata al ministro Franceschini, ma soprattutto sono accuse infamanti, a mio avviso gravi, che voglio stigmatizzare. È stato detto, infatti, che il ministro Franceschini avrebbe costruito tutta la sua carriera politica politica su uno scambio di favori, in relazione a scambi di interessi personali. Penso che questa cosa sia grave: non è una giustificazione il fatto che questo avvenga quando le telecamere possono dare più risalto; resta comunque e sempre, sia quando ci sono le telecamere,

desidero semplicemente far presente che non ho associato, come dice il collega, la carriera del Ministro a quella situazione. Ho detto che solo un Paese in cui ci sono una cronica mediocrità

da alcune settimane i viticoltori di Cirò, nel crotonese, territorio di antichissima tradizione vitivinicola, hanno lanciato l'allarme riguardo al Parco eolico denominato Timpe di Muzzunetti, che dovrebbe prevedere pale alte 200 metri nel cuore dei vigneti della DOC Cirò, a pochi passi dal mare, con impatto gravissimo sulla pianura del Fego e sulla valle del grazie l'ultima, nel 2018, permette di installare quattro aerogeneratori entro il 2021. Orbene, i tre parchi eolici già esistenti hanno inferto una grave ferita al territorio a Nord del Neto, punteggiato anche da pale isolate, sparse senza regole, e da mostri generati da un'edilizia incontrollata che suggella con il non finito il disordine urbanistico e l'incapacità di immaginare modelli di sviluppo che non prevedano l'utilizzo del cemento e il consumo di suolo. A fronte dell'ennesimo attentato al territorio, però, c'è stata una sollevazione della comunità cirotana, solidale con i viticoltori, perché conscia dei gravi rischi per le 50 cantine attive e per la fiorente economia del territorio, dove la crescente attività enoturistica nella qualità del paesaggio è un fondamentale elemento di attrazione, oltre alla qualità organolettica dei vini. I viticoltori non chiedono che il rispetto delle leggi già esistenti, signor Presidente: il quadro territoriale regionale paesaggistico (QTRP) del 2016, le linee guida nazionali sulle energie rinnovabili, l'articolo 9 della Costituzione e dunque il codice dei beni culturali del paesaggio, la normativa nazionale e regionale che regolamenta l'energia eolica in contesti riconosciuti di agricoltura di pregio, di paesaggi agrari consolidati e di produzioni agroalimentari di qualità. Proprio ieri il Consiglio regionale calabrese e quello comunale di Cirò Marina hanno preso posizione contro la realizzazione del parco eolico. Mi compiaccio per queste prese di posizione, ma l'attenzione deve restare massima e gli orientamenti espressi devono tradursi in atti concreti per la definitiva tutela dei distretti di pregio. In un territorio che vede ancora oggi tanti giovani emigrare, lo slancio di fiducia di chi vuole restare, pur tra mille difficoltà, per amore della propria terra, non sia umiliato da interessi privati che, oltre a una irrimediabile devastazione, null'altro lasceranno al territorio. Signor Presidente, vorrei tornare sulla questione della continuità territoriale. Come avevo già illustrato in un precedente intervento sul decreto-legge n. 45 del 2021 sui trasporti e le grandi navi, di gara svolto per garantire i collegamenti tra Arbatax e la terraferma, nella linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, è andato deserto. Il collegamento con l'Ogliastra è garantito per il mese di giugno e, da notizie stampa, apprendiamo che a luglio non ci sarà più. Invito pertanto la Presidenza a sollecitare una risposta all'interrogazione n. 4-05288 che abbiamo presentato per capire quali siano le reali intenzioni del Governo, se davvero intende tenere parte della Sardegna isolata dall'Italia, oppure se pensa che il collegamento con Cagliari sia sufficiente per assicurare la continuità territoriale navale nella linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, che, saltando Arbatax, diventerebbe Civitavecchia-Cagliari. Il Porto di Arbatax verrebbe tagliato fuori dai collegamenti marittimi di continuità territoriale, con la perdita di un'importante attività portuale e di posti di lavoro che attualmente vengono occupati.

Peraltro, è una spesa che va messa a regime per un servizio continuativo di continuità territoriale. Confido in una pronta risposta dal Governo per trovare una soluzione definitiva al problema.

Eppure il presidente Musumeci era stato avvisato del rischio saturazione di quel sito e della necessità di conferire fuori dall'isola, come da avviso pubblico bandito dal Dipartimento acqua e rifiuti, a conferma del fallimento delle politiche della sua Giunta, che verrà pagato a caro prezzo dai siciliani. La discarica di Lentini, oggi in amministrazione controllata, è stata gestita da Antonino e Salvatore Leonardi, rinviati a giudizio lo scorso 21 dicembre con l'accusa di aver creato un sistema di illecito smaltimento di rifiuti provenienti da oltre duecento Comuni siciliani, finalizzato all'esclusivo perseguimento di utili attraverso convenzioni con gli enti locali. Nessuna emergenza improvvisa, quindi, nessuna crisi delle ultime settimane. Il tanto decantato piano dei rifiuti non è servito a nulla. Basti pensare che, per ovviare all'attuale situazione, il Presidente della Regione Sicilia nei giorni scorsi avrebbe rispolverato l'idea dannosa e obsoleta di ricorrere agli inceneritori. Al contempo, si insiste sull'utilizzo delle discariche già esistenti, come quella di Cozzo Vuturo, nell'ennese, un impianto che, come denunciamo da anni, ha già mostrato i suoi limiti, dai rischi per l'ambiente a quelli per la salute dei cittadini di Enna e Calascibetta, grazie a tutti finanziato interamente con risorse pubbliche, che risolverebbe i problemi del trattamento dei rifiuti organici di un'intera provincia, possa essere stato svenduto per ripianare i debiti dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) di Enna, che ammontano a oltre 200 milioni, risultato di una scellerata gestione clientelare da parte della politica locale. Il caso ennese è solo l'esempio a me più vicino di come la questione rifiuti sia stata affrontata senza una visione di insieme. In Sicilia non occorrono inceneritori, ma piuttosto puntare all'obiettivo europeo del 65 per cento di raccolta differenziata e del 10 per cento come soglia massima da inviare in discarica. Vanno incentivati sempre più i comportamenti virtuosi in linea con i principi dell'economia circolare. Infine, occorre potenziare la rete di raccolta differenziata attraverso la creazione di *hub* dedicati al recupero dei rifiuti plastici e tessili, come previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasformando un problema in un'occasione di sviluppo, creando posti di lavoro e ponendo la Sicilia all'avanguardia nel settore del recupero. La transizione ecologica passa anche attraverso queste buone pratiche.

che hanno riversato alla foce di quello che era il biondo fiume tonnellate di rifiuti, che trasformano un paesaggio unico e suggestivo in un ambiente di degrado e pericoloso. Nonostante i periodici interventi di polizia a carico delle amministrazioni locali, i risultati sono veramente limitati, sia nel tempo sia nella quantità di rifiuti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

La seduta è tolta